Signor Presidente, onorevoli senatori, l'omicidio di Giulio Regeni ha scosso la nostre coscienze e il Paese intero, perché è stata troncata la vita di un giovane italiano esemplare, dottorando a Cambridge e ricercatore alla American University del Cairo, per il modo in cui è stato atrocemente torturato e ucciso e per la lezione di compostezza e di dignità che hanno dato i suoi genitori. Nell'informativa di oggi il Governo darà le valutazioni aggiornate sulla vicenda anche alla vigilia di importanti incontri che potrebbero essere decisivi per gli sviluppi delle indagini. A questo fine, credo sia importante che il Parlamento faccia sentire la propria voce unitaria. Come è noto, Giulio Regeni scomparve la sera del 25 gennaio al Cairo e il nostro ambasciatore, nei giorni seguenti, si attivò immediatamente, avendo colloqui con il Vice Ministro degli affari esteri, con la Consigliera per la sicurezza nazionale del Presidente e con il Ministro dell'interno. Io stesso, in quei giorni chiesi al mio omologo, il Ministro degli affari esteri egiziano, di attivarsi in tutti i modi possibili per scoprire le ragioni di quella scomparsa. Purtroppo il corpo di Giulio Regeni fu poi ritrovato il 3 febbraio. Dopo avere parlato con la madre, la signora Paola, che nel nel frattempo era arrivata al Cairo, diedi immediate istruzioni per chiedere formalmente, con una nota verbale, il rientro della salma in Italia e la partecipazione italiana alle indagini che sarebbero iniziate e, contemporaneamente, per convocare immediatamente l'ambasciatore egiziano al fine di esprimere Lo stesso giorno - parliamo del 4 febbraio - il presidente egiziano al-Sisi comunicava al Presidente del Consiglio l'assenso dell'Egitto all'arrivo del *team* italiano, che in effetti arrivò al Cairo due o tre giorni dopo il ritrovamento del corpo di Giulio Regeni. La posizione del Governo nei colloqui con le nostre controparti in Parlamento e in ogni sede è stata subito molto chiara. La riassumo utilizzando le parole del Presidente del Consiglio: ci fermeremo solo quando troveremo la verità, quella vera e non quella di comodo. Il fatto che l'Egitto sia un Paese chiave nella regione e che sia senz'altro un nostro alleato importante nel contrasto al terrorismo non è mai stato considerato un ostacolo, ma semmai deve essere considerato un incentivo a questa determinazione nel ricercare la verità. Allo stesso modo, quando poniamo il tema del rispetto dei diritti umani in Egitto, non lo facciamo certo per minare la stabilità di quel Paese; lo facciamo piuttosto, al contrario, per consolidare quella stabilità. Dopo una prima fase informativa, la collaborazione tra il nostro *team* investigativo e le Autorità egiziane, con il passare delle settimane, si è rivelata generica ed insufficiente. Per questo, a fine febbraio, ho anticipato al Ministro degli affari esteri del Cairo una nota verbale in cui il nostro ambasciatore ha poi formulato richieste molto precise e circostanziate, circa materiali che fanno parte dell'attività inquirente delle autorità egiziane (cinque tipologie diverse di materiale). Il 2 marzo, in seguito a questa nota verbale, un *dossier* di 91 pagine è stato consegnato alla nostra ambasciata e da noi immediatamente trasmesso alla procura della Repubblica di Roma, che nel frattempo aveva aperto un fascicolo di indagine. Non spetta a me entrare nel merito di questi documenti, e comunque non certo nei dettagli, ma la procura ha chiarito che questo *dossier* era certamente carente in generale e, in particolare, mancava di almeno due dei cinque capitoli di materiale richiesti dalla nostra nota verbale, quelli relativi al traffico di cella del telefono di Giulio Regeni e quelli relativi agli eventuali video della metropolitana del Cairo, nei pressi della quale potrebbe essere accaduto il sequestro del nostro concittadino. Devo dire che ulteriori difficoltà a questa collaborazione sono giunte poi dall'accavallarsi di notizie e versioni più o meno ufficiali o semiufficiali, smentite e verità di comodo che in questi ultimi due mesi sono circolate con troppa frequenza e quasi sempre al di fuori dei canali investigativi, peraltro istituiti tra Italia ed Egitto e tra le nostre autorità autorità inquirenti: dalla teoria dell'azione criminale volta a minare i rapporti tra i due Paesi (che certamente può essere un contesto, ma non è una risultanza investigativa), alle voci su Giulio Regeni informatore di questa o quella *intelligence*. Certamente questo non ha contribuito all'efficienza della nostra collaborazione. A metà marzo, la visita del procuratore della Repubblica Pignatone e del sostituto Colaiocco al Cairo ha rimesso questa collaborazione nei binari giusti. In quegli stessi giorni, come ricorderete, il Presidente egiziano al-Sisi ha dichiarato, in interviste rilasciate alla stampa italiana, di voler portare avanti fino in fondo l'attività di ricerca della verità. Tuttavia, dieci giorni dopo, il 24 marzo, il nostro *team* investigativo è stato convocato a tarda sera al Cairo per un *briefing* delle autorità investigative egiziane relativo all'uccisione di un gruppo di cinque criminali dediti a rapinare o a sequestrare cittadini stranieri spacciandosi per poliziotti. Nel *briefing* è stato detto ai nostri investigatori che nell'abitazione del capo di questo gruppo di criminali era stata trovata una borsa contenente, tra altro, il passaporto e i tesserini universitari di Giulio Regeni. Questo è apparso come un ulteriore e ancor più grave tentativo di accreditare una verità di comodo e la reazione italiana è stata ferma e immediata. Sia il Governo che la procura della Repubblica di Roma, con i rispettivi canali, hanno subito chiarito che non avremmo accettato questa come la conclusione dell'indagine. La famiglia, come sapete, ha reagito pubblicamente e con forza. Nei giorni successivi diversi esponenti del Governo egiziano, smentendo smentendo di fatto la teoria che faceva risalire a quel gruppo di criminali l'omicidio di Giulio Regeni, hanno chiarito che le indagini sono ancora in corso e di questo noi prendiamo atto, fino al punto - e lo voglio segnalare - che due giorni fa il principale quotidiano egiziano, «Al-Ahram», in un editoriale del suo direttore, si è spinto a chiedere pubblicamente allo Stato di individuare e di punire i responsabili. Questa è la situazione ad oggi. A questo punto, onorevoli senatori, credo sia legittimo e, anzi, doveroso chiedersi se la fermezza della reazione del Governo, della magistratura, della famiglia e dell'Italia intera potranno riaprire un canale di piena collaborazione; il canale, peraltro, assicurato dallo stesso presidente al-Sisi. Lo capiremo a partire dall'incontro tra gli inquirenti, che è previsto per giovedì e venerdì di questa settimana e a cui parteciperanno cinque tra magistrati e investigatori egiziani. magistrati e investigatori egiziani. Cosa vuol dire ristabilire un canale di piena collaborazione? Vuol dire, innanzitutto, acquisire la documentazione mancante, quella che sappiamo esistere e che abbiamo formalmente richiesto; vuol dire non accreditare verità distorte o di comodo; vuol dire accertare chi fossero i responsabili della probabile messa sotto osservazione di Giulio Regeni nel periodo precedente alla sua scomparsa; vuol dire accettare l'idea che l'attività investigativa possa vedere un ruolo più attivo degli investigatori italiani, ovviamente sotto la responsabilità degli inquirenti egiziani, come previsto dalla legge. Sarà anzitutto la procura della Repubblica a valutare se questo cambio di marcia si delinei. Lo capiremo e lo valuteremo insieme nei prossimi giorni, senza inseguire oggi questa o quella voce, questa o quella anticipazione giornalistica.

se questo cambio di marcia non ci sarà, il Governo è pronto a reagire adottando misure immediate e proporzionali e il Parlamento ne sarà tempestivamente informato. Onorevoli colleghi, ho sentito richiamare - più o meno correttamente, ma spesso - in questi giorni, attorno a questa vicenda terribile, la ragione di Stato. Fatemi, allora, dire ancora una volta che cosa ci impone, in un caso come questo, la ragione di Stato. Ci impone di difendere, fino in fondo e nei confronti di chiunque, la memoria di Giulio Regeni, nel cui barbaro assassinio la madre ha visto palesarsi, come ha detto, «tutto il male del mondo». È dunque per ragione di Stato che pretendiamo la verità, è per ragione di Stato che non accetteremo verità fabbricate ad arte, è per ragione di Stato che non ci rassegneremo all'oblio di questa vicenda ed è soprattutto per ragione di Stato che non consentiremo che venga calpestata la dignità del nostro Paese. *(Applausi

ma, in tutte le occasioni in cui il nostro Paese è esposto sul piano dei rapporti internazionali, ci piace e ci piacerebbe continuare a non essere e non sentirci all'opposizione. In questa drammatica vicenda credo che possiamo dare atto non solo stamattina, ma già da quei terribili giorni tra il 25 gennaio e il 3 febbraio

dignità. Come lei auspicava stamattina, possiamo auspicare anche noi di essere alla vigilia - mi pare tra giovedì e sabato prossimi - di sviluppi che potranno rivelarsi decisivi per le indagini. Se così fosse, vorrebbe dire che quella linea da lei interpretata di istituire subito canali investigativi italo-egiziani era una via giusta, ferma e dignitosa, la quale ha dato i suoi risultati, a prescindere a prescindere dalle incompletezze della documentazione, dall'accreditamento fantasioso di versioni occasionali e dall'inseguimento di questa o quella anticipazione giornalistica.

ha ricordato anche lei, signor Ministro - sia del dottor Pignatone, sia del suo vice, dottor Colaiocco. Francamente ci incuriosisce e appassiona molto meno il dibattito in seno ad alcuni magistrati o ex magistrati in cerca di gloria. Ve ne è uno francamente squallido e penso al dibattito di stamattina tra il procuratore Spataro di Torino e il dottor Ingroia, su quello che compete alla magistratura nei rapporti internazionali. Le nostre ragioni di lealtà allo Stato democratico implicano che le rappresentanze diplomatiche all'estero e non abbiamo che da esprimere stima per il comportamento tenuto dal nostro ambasciatore a Il Cairo - sono certamente rappresentanze di Governo, ma anche della statualità nazionale. Quindi, questo dibattito scomposto avviato stamattina su un quotidiano da Spataro e Ingroia, non ci appassiona minimamente. Attendiamo con la sua stessa fiducia per il fine settimana, augurandoci che da esso possa salutarsi il ritrovamento, ammesso che lo si fosse mai smarrito, di un rapporto di piena collaborazione. Altrimenti, ci rimettiamo a quelle che stamattina lei, signor Ministro, ha definito misure immediate e proporzionate. Non vogliamo saperne, né vogliamo indicare di più,

non intendiamo minimamente strumentalizzare o servirci della memoria di Giulio Regeni per muovere con lui, come strumento, il processo agli sforzi del generale al-Sisi per far ritrovare al suo Paese calma, compostezza e tranquillità. È importante legare la calma e la compostezza dei rapporti tra l'Italia e l'Egitto al non verificarsi casi di torture, così frequenti in Egitto in passato, così accreditati dalla genia dei cosiddetti Fratelli musulmani che oggi - loro sì - strumentalmente si servono della memoria martoriata di Giulio Regeni e del dolore dei suoi familiari per un contenzioso di politica interna con il generale al-Sisi. Ecco perché abbiamo ascoltato con molto rispetto e ci atteniamo alle sue

Signor Ministro, onestamente le dobbiamo dire che un po' di delusione c'è sempre quando

un nostro rispettoso e affettuoso saluto alla famiglia di Regeni e alla madre, a quella donna che ci ha dato una grandissima lezione di dignità. Quella madre, però, nel suo argomentare ha lanciato anche un messaggio forte, a noi e a voi governativi *in primis*: dobbiamo dare delle risposte al Paese. madre ha detto che, se ci saranno ancora ritardi, confida in una risposta forte. Lei, Ministro, ha detto che ci sarà e noi vorremo capire come, quando e se. oggi: il recupero di effetti personali di Regeni in un appartamento attribuito ad una banda di criminali che, camuffati da poliziotti, sarebbero dediti al sequestro di persone e a rapine.

sul corpo straziato di Regeni non potevano che essere opera di persone esperte e addestrate alla tortura.

che tutti noi chiediamo e vogliamo e che voi del Governo dite di volere perseguire. Però, Ministro, guardiamo il quadro complessivo: qui abbiamo un ragazzo che è incaricato da un'università inglese di andare a fare ricerca in ambiti estremamente sensibili e in un Paese del quale tutti conoscono l'instabilità.

i Servizi possono anche rinunciare a mandare agenti sotto copertura e affidare addirittura un incarico ad un altro istituto, in questo caso un istituto

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il caso di Giulio Regeni rappresenta una pagina drammatica sulla quale l'Italia, davvero senza distinzioni di parte, chiede ed esige la verità. Con la morte di Giulio Regeni è stata spezzata una giovane vita e anche, allo stesso tempo, un ideale: l'ideale di una gioventù che viaggia, studia all'estero e va a conoscere nuove culture. Sullo scenario internazionale, come l'attualità spesso drammatica insegna, e soprattutto (per restare vicino a casa nostra) nella regione del Mediterraneo viviamo momenti difficili e complessi: la conflittualità e la tensione sono alte. I giovani - lo dico davvero senza alcuna retorica - sono la nostra speranza per un futuro migliore. Anche per questo la tragedia di Giulio Regeni, la sua morte arrivata al culmine di torture e sofferenza, è un colpo al cuore non solo dell'Italia. Lo dimostra la grande e sentita eco che la morte di Giulio Regeni ha avuto all'estero. A questa ondata di commozione, ancora una volta, il Gruppo parlamentare a cui appartengo desidera associarsi. Siamo vicini alla famiglia di Giulio Regeni e, idealmente, a tutti quanti - anche in Egitto - invocano una verità finale e credibile su quanto avvenuto. Sono passati oltre due mesi da quel drammatico 3 febbraio e a parere del nostro Gruppo l'incessante richiesta da parte del Governo italiano nei confronti delle autorità egiziane perché la famiglia Regeni - e con essa l'intero Paese - sappia cosa è accaduto, va nella giusta direzione. Attendiamo con ansia di conoscere gli esiti dell'incontro che, il 7 e l'8 aprile, vedrà impegnati gli investigatori italiani e gli inquirenti egiziani, guidati dall'assistente del procuratore generale egiziano. Al tempo stesso bisogna essere molto netti e sottolineare che la versione annunciata dalle autorità egiziane a fine marzo, come oggi il signor Ministro ci ha riportato, non ha convinto, né poteva convincere nessuno, così come non poteva minimamente darci sollievo. Non a caso lo stesso Governo egiziano ha successivamente fatto sapere - con il Ministro dell'interno - di non poter essere certo che Regeni sia stato ucciso da una banda specializzata nelle rapine agli stranieri, come ipotizzato invece dagli investigatori del Cairo. Secondo alcuni osservatori le parole del Ministro egiziano sono state un primo parziale segnale di ammissione da parte egiziana del fatto che la verità su Giulio Regeni sia in realtà diversa da quella annunciata in prima battuta. Non possiamo che attendere con attenzione gli sviluppi dell'inchiesta e, al tempo stesso, affermare con forza che il Parlamento italiano chiede a gran voce che tale inchiesta sia vera, completa e senza indugi: in una parola, che sia credibile. Qui non possiamo nasconderci il risvolto politico, che è della massima importanza, della vicenda Regeni. L'Italia, con realismo e concretezza, è stato tra i Paesi della comunità internazionale che hanno voluto dare fiducia, in modo chiaro ed espresso, al nuovo Governo egiziano del presidente al-Sisi. La fiducia data dall'Italia a tale Governo merita, da parte egiziana, di essere contraccambiata con risposte e un impegno nella soluzione del caso Regeni che siano all'insegna della chiarezza, della limpidezza e di un vero impegno nella ricerca della verità. Il nostro augurio è che quanto dichiarato pochi giorni fa dal Ministro degli affari esteri egiziano, che ha parlato di «determinazione e impegno totale del Governo egiziano e degli apparati di sicurezza a continuare gli sforzi per scoprire la verità», abbia un seguito concreto. Apprezziamo le dichiarazioni ufficiali di un Paese, che resta amico dell'Italia, come l'Egitto, ma ancora di più le apprezzeremo nel momento in cui emergerà tutta la verità. Una verità che non deve essere a tutti i costi, altrimenti ci saremmo accontentati della prima e poco credibile verità emersa. fa le ho inviato una lettera su di un incontro che la nostra delegazione all'Assemblea parlamentare del Mediterraneo ha avuto con il Presidente e una delegazione di parlamentari egiziani, che in quella occasione espresse grande cordoglio al Paese e alla famiglia per l'omicidio Regeni e, al tempo stesso, la fermezza del Parlamento egiziano a ricercare "la vera verità". Signor Ministro, come abbiamo avuto modo di esprimere ancora poche settimane fa, sempre in quest'Aula, in occasione della sua informativa sulla Libia le vicende mediorientali e nordafricane sono motivo di preoccupazione. In quell'occasione parlammo in modo diffuso dell'instabilità e del caos presenti in Libia. La situazione dell'Egitto è certamente diversa, ma va certo vista nel più ampio contesto di un'area che vive anni di massima tensione. La cosiddetta Primavera araba dell'Egitto, come avvenuto in altre realtà del Nord Africa, non ha realizzato le promesse di rinnovamento che alcuni avevano intravisto. Le complesse vicende egiziane seguite alla caduta di Mubarak, avvenuta nel 2011, sono e saranno anche nei prossimi anni oggetto di analisi e discussione. Di fatto, con il Governo al-Sisi si sono poste le basi per cercare di dare a quel Paese, grande, popoloso e straordinariamente strategico per i sempre labili equilibri di quella regione e in generale del mondo arabo, un minimo di stabilità, anche per gli investimenti esteri. La linea politica tenuta dall'Italia è giusta e, a nostro parere, va portata avanti ma, ancora una volta, ciò non può farci desistere dall'esigere la verità su Giulio Regeni. In un'intervista pubblicata alcuni giorni fa sul «Corriere della sera», lei, signor Ministro, ha affermato che l'Italia sarebbe pronta a trarre le opportune conseguenze qualora dall'Egitto non arrivassero risposte credibili. Oggi lo ha ripetuto in quest'Aula. Attendiamo con attenzione, come detto in precedenza, gli esiti del vertice investigativo dei prossimi giorni, ma avendo ben chiaro che tutta l'Italia vuole verità e giustizia per Giulio Regeni e che dobbiamo essere fermissimi nel far comprendere alla controparte egiziana che, appunto, l'Italia è davvero determinata nella richiesta di verità. Ecco perché oggi le sue sono state parole di chiarezza che noi condividiamo *in toto*.

la sua informativa condividendone i contenuti, appoggiando la linea che il Governo sta seguendo sin dal primo momento e sostenendo il gravoso compito di ordine diplomatico e giudiziario che accompagnerà i prossimi mesi. Certo, la tematica è estremamente delicata perché inerisce alla politica internazionale. La vicenda di Giulio Regeni, appena ventottenne, dottorando di ricerca dell'American University e laureto e ricercatore alla Cambridge University è la testimonianza di come in alcune zone del mondo, nel vicino Egitto evidentemente, non c'è spazio, non c'è luogo, non c'è possibilità perché si possano affermare in maniera inequivocabili i diritti fondamentali dell'uomo. Non solo, ma il suo intervento ha richiamato - a me sembra - due parole chiave:

Lei ha opportunamente sottolineato, in una formulazione estremamente corretta e condivisa (se lei mi permette di usare questa espressione di consenso), che non è in discussione il ruolo dell'Egitto per la stabilità di una regione particolarmente tormentata e al centro di tante tensioni internazionali, non è in dubbio il sostegno a un Paese fortemente impegnato contro la minaccia terroristica, ma è in discussione la fine atroce di un nostro connazionale, torturato e barbaramente ucciso. Su questa vicenda, il Governo e il Presidente della Repubblica ancor più hanno chiesto immediatamente che si arrivasse alla verità e alla punizione dei colpevoli. Le circostanze di queste settimane, di questi due mesi passati molto rapidamente, non hanno evidenziato a tutt'oggi alcuna verità che possa essere plausibile; solamente delle pseudoverità che lei giustamente ha richiamato, direttamente e indirettamente, essere forme un po' originali di depistaggio, alla ricerca di una verità che, a me sembra, richiederà ancora molto, molto tempo. La sua posizione, la posizione del Governo, è stata immediatamente molto ferma. A me sembra, signor ministro Gentiloni, che l'impegno del Governo non sia più soltanto quello del Governo italiano, possa essere di monito a livello internazionale, perché la vicenda di Giulio Regeni che ha colpito l'Italia ha un respiro internazionale. Gli ultimi dati riportati da Amnesty International parlano di 88 casi di così definite sparizioni dall'inizio del 2016, cioè appena quattro mesi orsono, di cui otto casi di morte accertata. Altre organizzazioni non governative hanno evidenziato negli ultimi otto mesi ben 533 sparizioni forzate (così definite), il che vuole dire sparizioni che richiamano vicende oscure della storia internazionale.

lei giustamente ha richiamato in un passaggio che il Parlamento si possa esprimere in maniera univoca. Non c'è su queste tematiche alcuna differenza tra maggioranza e minoranza, maggioranza e opposizione. Qui è in discussione la dignità dello Stato, ma soprattutto la libertà di pensiero di giovani ricercatori, di persone come Giulio Regeni, che rappresentano una unicità della qualità del pensiero dei nostri concittadini. Vorrei terminare questo mio breve intervento, signor Ministro, richiamando un'espressione di Ferdinando Camon, che ha scritto oggi un editoriale su un quotidiano che

rilevanza. Sullo scenario internazionale, la tragedia di Giulio Regeni è l'attenzione che il mondo internazionale ha verso il percorso di maturazione democratica dell'Egitto, che dovrebbe essere uno dei Paesi

non può che generare una grande preoccupazione e una notevole attenzione, tant'è che questo viene testimoniato dall'interessamento delle grandi potenze sul caso particolare. Sullo scenario nazionale tale elemento si sovrappone

italiano come noi: egli finisce per essere fratello, figlio di tutte le madri, e proprio con questa considerazione dovremmo fare tutti tutti molta più attenzione a trattare il caso con una maggiore prudenza. Cosa si vuole

una rilevanza notevole ai lati oscuri, dimenticando che il nostro è un Paese che rispetto agli altri in tanti decenni non è riuscito a fare chiarezza su fatti che invece avrebbe avuto il dovere di chiarire. Un Paese, il nostro, di cui ancora oggi si parla - della strage di Ustica, di piazza Fontana, di Brescia, degli omicidi eccellenti - senza riuscire ad avere

da questa immaturità tutta italiana e a fare quello che per gran parte sta facendo, e cioè essere attento alle ragioni dell'Italia, ma ancor più alle ragioni dell'individuo quale che sia (italiano, inglese, siriano, americano) siriano, americano) perché in nessuna parte del mondo possa succedere quello che è avvenuto al Cairo. In questo senso credo che il Governo stia facendo la sua parte, e ancora di più la sta facendo abbastanza bene.

che per l'Italia è stato raggiunto l'estremo limite della pazienza. Abbiamo perso il conto delle bugie, delle infinite versioni di comodo, degli sgangherati tentativi di depistaggio che cercano di nascondere quello che non può essere nascosto, e che io credo sia davvero evidente a tutti, non solo in quest'Aula ma nell'intero Paese. Giulio Regeni, un ragazzo di ventotto anni che intrecciava un brillante impegno di studioso con la passione civile e democratica, è stato barbaramente torturato e ucciso

Sinora il Governo egiziano si è prodigato con ogni mezzo non per raggiungere questo obiettivo, ma per impedirlo. Ognuna delle bugie dette in questi mesi - e poi ritrattata soltanto per dirne una nuova - rappresenta un insulto alla memoria di Giulio Regeni ai suoi genitori, che hanno avuto la dignità e la forza di essere qui con noi proprio nell'importante conferenza stampa organizzata dalla Commissione diritti umani. In definitiva, un'offesa alla dignità del popolo italiano e finanche delle sue istituzioni democratiche. Se anche l'incontro tra gli inviati egiziani e il procuratore Pignatone si concluderà con un nulla di fatto diventerà - crediamo - inevitabile una drastica iniziativa del Governo italiano, che avrebbe già dovuto agire con più determinazione di fronte alla evidente e palese mancanza di collaborazione, e anzi del metodico sabotaggio da parte delle autorità egiziane. Per noi questa è davvero l'ultima scadenza. Sappiamo tutti perché ciò non è stato fatto finora e quali considerazioni suggeriscano di evitare un conflitto diplomatico. Non vogliamo nemmeno sottovalutare l'interscambio commerciale con l'Egitto, per esempio, o anche la possibilità di sfruttare il giacimento di gas scoperto dall'ENI a largo di Zohr, che ha un ovvio valore strategico, né vogliamo, naturalmente, dimenticare il ruolo che può avere l'Egitto nel fronteggiare il crescente fondamentalismo islamico, ma ci sono momenti nei quali un Paese è chiamato a scegliere tra la difesa dei principi che proclama inviolabili e i calcoli della *realpolitik*. Ed è da questa scelta che dipendono la sua identità, la sua dignità e, alla lunga, anche la sua credibilità internazionale. Questo è vero non solo per il caso che ci tocca da vicino di Giulio Regeni. Tra le tante bugie che abbiamo dovuto ascoltare in questi mesi, quella pronunciata pochi giorni fa dal Ministro degli affari esteri egiziano è davvero drammaticamente clamorosa: l'uccisione di Regeni, ha detto, è un atto isolato. Non è vero; non è così. Negli ultimi otto mesi 533 persone sono state rapite dai Servizi di sicurezza egiziani. Di 369 di quelle persone non si sa più niente. Chiamiamoli con il loro nome: sono *desaparecido*, vittime di un regime non diverso da quelli criminali di Videla in Argentina o di Pinochet in Cile. Avere appoggiato quei regimi in nome della *realpolitik* è stato per molte potenze occidentali uno dei capitoli più vergognosi della guerra fredda ed è stato anche un errore strategico per il quale l'Occidente continua a pagare durissimi prezzi. Non si può rifare oggi quello stesso tragico sbaglio in nome della guerra al Daesh o dell'emergenza profughi. Il nemico del proprio nemico non può essere sempre e comunque un amico. Non si possono chiudere gli occhi sulle violazioni continue dei diritti umani che a parole, peraltro, tutti quanti noi proclamiamo sacri. Abbiamo davvero tutti i motivi per credere che Giulio Regeni sia stato torturato e ucciso proprio perché indagava e studiava su quelle violazioni di diritti umani, sociali e politici che nell'Egitto di al-Sisi sono all'ordine del giorno. Combattere quelle violazioni senza farci distrarre da considerazioni reali, ma di ben più piccolo cabotaggio è ciò che tutti noi dobbiamo alla sua memoria, alla dignità democratica dell'Italia e, infine, a noi stessi. Verità e giustizia per Giulio Regeni!

nei giorni scorsi, le parole del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio e, questa mattina, le parole del nostro Ministro degli affari Penso che se avessimo potuto rinunciare a questo dibattito, veramente nelle parole del Ministro degli affari esteri si sarebbe potuto ritrovare tutto il Parlamento, ha espresso parole equilibrate e nette che hanno rassicurato il Senato sul fatto che noi non siamo un Paese barzelletta e non accetteremo, in questa vicenda, le tante bugie e verità di comodo che hanno cercato di propinarci in queste drammatiche settimane.

In questo momento parliamo di una vicenda drammatica che riguarda una splendida famiglia italiana - i genitori, la sorella e Giulio - e di quello che sono nell'immagine degli italiani e nella nostra, nostra, di quel piccolo paese che, pieno di dignità, ha ricordato Giulio, e di una comunità internazionale di universitari che sta dietro agli sforzi di un ricercatore esemplare come tanti nostri figli che sono in giro per il mondo. Bene. Però la misura e la fermezza del nostro Ministro degli affari esteri valgono di più, onorevoli senatori, perché il Ministro degli affari esteri sa che che cosa c'è dietro a questa vicenda, conosce cioè il quadro che un responsabile politico non può far finta di non vedere o dimenticare. Senatore De Cristofaro, conosco il suo *pathos*, so quanto sia autentico e sincero. Nei giorni scorsi mi sono trovato dalla Tunisia a parlare di Giulio Regeni ad «Al Jazeera» e a metà della trasmissione cui ho partecipato ho capito sinceramente che da essa traspariva non solo la giusta indignazione, che condividevo,

che lavorano in questo momento probabilmente non avendo la preoccupazione che abbiamo noi (autentica, dal primo all'ultimo in quest'Assemblea) di Giulio Regeni, ma preoccupazioni diverse, coincidenti con gli interessi che si muovono tra il Golfo e il Mediterraneo

e non possiamo credere alla barzelletta che Haftar combatte contro il governo dell'ONU se non ha alle spalle qualcosa di consistente che lo tiene in piedi (apro e chiudo la parentesi). Stiamo attenti in questa vicenda a non spostarci da una rigorosissima e consistente posizione

che per difendere la memoria di Giulio Regeni il Governo è pronto ad adottare misure proporzionate e adeguate se non ci sarà la collaborazione. A me bastano queste parole; mi bastano sinceramente perché capisco che mai come in questo caso il Parlamento è in sintonia con il Governo e che il Governo non accetta di essere preso in giro. Fino a oggi abbiamo ritenuto che la nostra *partnership* privilegiata con l'Egitto non fosse un problema, ma fosse la chiave della soluzione e vogliamo continuare a pensare questo. Ma con i nostri amici egiziani dobbiamo essere molto chiari e mettere le carte in tavola, perché se abbiamo ritenuto questo fino ad ora probabilmente loro hanno pensato qualcosa di diverso, perché ci sono state somministrate troppe bugie, in modo ripetuto e sistematico, per non farci pensare male, a partire dalle ricostruzioni nel momento immediatamente successivo al ritrovamento del corpo di Giulio, fino alle ultime, al misterioso ritrovamento dei documenti di Giulio Regeni in una circostanza che, peraltro, è la prova provata di come all'interno del regime ci siano delle responsabilità. Questa è la questione.

e lotte di potere all'interno del sistema egiziano che devono venire alla luce e che al-Sisi deve far venire alla luce. Non è in il decoro di una Nazione come l'Italia, ma è anche quella credibilità minimale (non dico quella credibilità, ma, ripeto, quella credibilità minimale) che l'Egitto devo conquistarsi sul campo. Infatti per noi la verità più terribile che può esserci disvelata, la più terribile per questo ragazzo e per la sua famiglia, è preferibile alle bugie. Noi dobbiamo essere disponibili ad accettare anche il più drammatico dei verdetti che ha un requisito non banale, quello di essere vero, di essere verità, perché questo è quello che il Governo italiano, il nostro Parlamento e il nostro popolo vogliono in una vicenda che chiama in causa il decoro nazionale. Dunque la ragion di Stato, per quanto ci riguarda, in questo caso non è in conflitto con la ricerca della verità. La ragion di Stato ci porta a vedere - questo sì, ma è un'altra pagina non confondibile - che l'Egitto è a uno snodo fondamentale, che è un *partner* decisivo per un minimo di stabilità nel Mediterraneo e che noi dobbiamo lavorare, proprio con l'autorevolezza che il Governo sta dimostrando, per stabilizzare questa area martoriata del Mediterraneo e del Nord Africa. infine rivolgere un ringraziamento all'ambasciatore Massari, che opera in Egitto e che è la dimostrazione di come i diplomatici italiani, nella stragrande maggioranza, sono persone che servono con lealtà, decoro ed intelligenza il loro Paese. *(M5S)*. Signor Presidente, purtroppo devo contestare quanto è stato affermato questa mattina in quest'Aula: abbiamo ascoltato parole che ci lasciano sinceramente allibiti. Caro presidente Casini, quel giorno i genitori di Giulio Regeni ci hanno chiesto delle cose: ci hanno chiesto principalmente di fare il nostro lavoro significa, anche per noi, dire e raccontare al Paese la verità. Quindi rispondo anche a qualcuno che ci ha attaccato ed indico il ministro Gentiloni presente qui in Aula. Le vostre mani in questo momento - e, quando dico "vostre", mi riferisco maggioranza, al PD in particolare - sono sporche e sono colorate di rosso e di nero. Una mano è sporca di nero perché è sporca di petrolio, l'altra di rosso perché è sporca di sangue. Noi siamo presenti in Aula, ma i nostri colleghi sono sul territorio e stanno combattendo un conflitto. Questo conflitto è un conflitto di interessi nella vostra battaglia, che perderete. *(M5S)*. Quello che posso dirvi è che il vostro è un Governo complice e vi spiego perché. Questo è l'elenco dei trattati internazionali che il nostro Governo ha firmato in materia di assistenza giudiziaria. L'abbiamo fatto soltanto con l'Algeria, il Libano, il Marocco e la Tunisia; se l'avessimo fatto anche con l'Egitto, ora il procuratore Pignatone potrebbe avere le mani più libere. Ma voi non lo fate!

Cociancich, Cirinnà, Fabbri: vergognatevi! Noi siamo sul territorio a combattere!

Vorrei sottolineare il fatto che, dietro a questa vicenda (è per questo che ho parlato di mani rosse e nere), la risoluzione del Parlamento europeo chiede una cosa molto semplice: la sospensione della fornitura di armi all'Egitto, per un motivo molto semplice.

e 500 prigionieri sono morti nelle carceri egiziane. È questo il Governo con il quale voi fate affari, per un totale di 5 miliardi di euro l'anno, ed è per questo motivo che siete complici! un'altra questione che non avete affrontato e di cui non hanno parlato né il ministro Gentiloni, né il presidente Casini: la relazione annuale sull'*impor**t‑export* di armi, che ogni anno il Governo dovrebbe presentare al Parlamento dov'è? Non ce n'è notizia neanche quest'anno. Sono queste le informazioni che ci dovete dare, sono queste le verità dietro le quali c'è anche il caso Regeni! Vogliamo parlare dell'Egitto? Questo è il motivo per cui voi siete totalmente inefficienti, perché l'Egitto è un nostro *partner* commerciale. Abbiamo affari con oltre

ritiene non soddisfacente la sua informativa. È per questo motivo che avevamo chiesto non una semplice informativa, ma delle comunicazioni. in quel caso, avremmo potuto presentare risoluzioni e mettere nero su bianco un voto da parte dell'Assemblea. La sua informativa non ci soddisfa;

signor Ministro, colleghi senatori, quella odierna è una pagina triste della nostra vita parlamentare: parliamo di un ragazzo italiano innocente, morto in circostanze oscure, circostanze oscure, sulle quali l'Italia intera e probabilmente non solo l'Italia chiedono ed esigono chiarezza. Credo che la chiarezza su quanto accaduto - che non è affatto scontato - sia interesse prima di tutto dello stesso Governo egiziano, che - voglio ricordarlo - è amico dell'Italia e dell'Occidente. Un Governo che sta svolgendo un compito essenziale nella lotta contro l'integralismo islamico e che per questo è malvisto da molti degli amici, dei fiancheggiatori e dei simpatizzanti, più o meno occulti, di Daesh, ovvero ISIS. L'Egitto - non dimentichiamolo - dopo la caduta di Mubarak, era caduto nelle mani della Fratellanza musulmana. Voglio solo ricordare in quest'Assemblea, come testimonianza, il motto dell'organizzazione dei Fratelli Musulmani recita: «Dio è il nostro obiettivo. Il profeta è il nostro capo. Il Corano è la nostra legge. Il *jihad* è la nostra via. Morire nella via di Dio è la nostra suprema speranza». Le sfide di libertà di piazza Tahrir, che tanto avevano emozionato gli occidentali, si erano presto trasformate (per via del tutto democratica, a dire il vero) in un regime teocratico, quello del presidente Morsi, che andava ogni giorno di più stringendo le sue maglie; un regime che stava spostando il peso politico e morale dell'Egitto dalla parte dei nemici dell'Occidente e della libertà. È una triste, ma frequente prassi nel mondo islamico che siano i militari i garanti della laicità dello Stato contro il clericalismo islamico. È accaduto per lungo periodo in Turchia, è accaduto in un passato non troppo lontano in Algeria e accade oggi in Egitto. Sappiamo bene che il Governo di al-Sisi non rispetta le regole democratiche come le intendiamo noi in Occidente. Sappiamo altrettanto bene che costituisce il modello di governo migliore possibile oggi, nelle condizioni storiche date, in Egitto. Una piena democrazia, come la intendiamo noi, è un processo da realizzare nel tempo, non una realtà da imporre dogmaticamente a un Paese in guerra. Questo è il contesto nel quale ho voluto inserire l'omicidio di Giulio Regeni. Oggi abbiamo ascoltato il Ministro. Signor Ministro, lei non ci ha dato grandi novità: la maggior parte delle informazioni che abbiamo sentito da lei le abbiamo ampiamente lette nei giornali in questi giorni. Ha parlato di un ruolo più attivo degli investigatori italiani, di un eventuale cambio di marcia; ha detto che non inseguiamo questa o quella voce giornalistica; ha anche detto che se il cambio di marcia non ci sarà si dovranno prendere misure adeguate e proporzionali, senza, però, specificare quali saranno queste misure adeguate e proporzionali. Ha specificato anche, a conclusione della sua comunicazione di oggi, che la ragione di Stato, in questo caso - e forse non solo in questo - impone solo di conoscere la verità, ovvero quello che è accaduto effettivamente a Giulio Regeni. Devo dire che l'unica novità che abbiamo appreso (ma anche questa è presente sui giornali) è che gli investigatori egiziani, invece di venire domani, come forse lei ha detto prima, arriveranno il 7 aprile nel nostro Paese. Quindi, cosa sia successo a Giulio Regeni noi oggi probabilmente non lo potevamo sapere. Ma non abbiamo nemmeno capito con quali strumenti si possa conoscere la verità. Non conosce la risposta lei, signor Ministro, non la conosciamo noi e non la conosce il Parlamento. Potrebbe essersi trattato di un atto di eccesso di zelo di qualche funzionario; potrebbe trattarsi di un errore di persona; potrebbe trattarsi di una provocazione di qualche ramo deviato dello Stato ai danni dello stesso Governo di al-Sisi.

una sfida globale che ci riguarda direttamente per la nostra collocazione geografica, la nostra vocazione storica e il ruolo simbolico di Roma come sede della tradizione classica su cui si basa il concetto stesso di Occidente e, naturalmente, come centro della cristianità. È una sfida in cui è fondamentale avere chiaro chi sono i nostri amici e quali sono i nostri nemici e in cui - naturalmente - è giusto chiedere ai nostri amici di aiutarci e capire cosa è successo davvero a un nostro connazionale e assicurare alla giustizia il responsabile di un delitto ancora più atroce perché senza senso e logica. Possiamo chiederlo e ottenerlo se dalla propaganda passiamo alla politica, alla diplomazia e alla collaborazione giudiziaria. Spero che, d'ora in poi, il Governo Renzi si muova in questa direzione.

non lo meritano i nostri connazionali in Italia e all'estero. Signor Presidente, signor Ministro, la ringraziamo per la sua informativa, che apprezziamo e condividiamo per l'equilibrio e la determinazione. Ci dispiace molto aver ascoltato le farneticanti parole del senatore Lucidi, davvero poco lucide

e chiedono che sia rimosso ogni ostacolo al raggiungimento della verità, ottenendo dalle autorità egiziane la doverosa collaborazione senza omissione e reticenze. Il Ministro ha parlato francamente oggi delle molte carenze e contraddizioni nelle posizioni tenute fin qui dall'Egitto. Per questo, è ora indispensabile che la verità emerga, tutta e completa, mettendo a disposizione tutte le carte e gli elementi dell'indagine. Lo dobbiamo alla memoria di Giulio Regeni, alla sua figura di intelligente e appassionato ricercatore, alla sua passione per lo studio e per la conoscenza. Lo dobbiamo alla famiglia di Giulio, al suo appello accorato perché l'oblio non cada mai su questa oscura e tragica vicenda. Vorrei qui ringraziare l'azione della Commissione per i diritti umani e del presidente Manconi, che ha dato la giusta cornice ed il risalto dovuto senatrice Bencini)* perché l'Italia non si dimentichi di un suo figlio generoso ed impegnato e ottenga la verità. Lo dobbiamo infine al nostro Paese e all'opinione pubblica internazionale, a cominciare da quella egiziana. Molti commentatori e testimoni dell'Egitto di oggi ci dicono che la morte violenta di Giulio Regeni non è un caso isolato in quel Paese, che i segnali di un uso ampio e incontrollato di forme di intimidazione, violenza e tortura sono molteplici e preoccupanti. L'Egitto svolge un ruolo strategico di cerniera nel Mediterraneo e nel Medioriente ed è importantissimo che giunga subito dalle sue autorità un messaggio vero di apertura, di collaborazione, di efficienza. Ci aspettiamo novità forti, credibili e decisive dal prossimo incontro tra i magistrati egiziani e quelli italiani. È il tempo adesso di indagini rigorose, condotte con aperta e trasparente collaborazione, spegnendo sul nascere i tentativi di depistaggio o di intorbidamento delle acque. L'Egitto è per l'Italia un importante alleato nella lotta al fondamentalismo e negli sforzi di stabilizzare la pace e la sicurezza nell'intera regione. Questo rapporto di amicizia consente un colloquio franco e diretto. Noi non accetteremo versioni accomodate o nascondimenti della verità. Proprio perché siamo Paesi vicini e amici, ne va del futuro delle nostre relazioni, per le quali la soluzione del caso Regeni è un vero e dirimente banco di prova. Noi non ci rassegneremo mai al dilemma: «o i diritti umani o i rapporti politico-commerciali». Questi due aspetti non sono scindibili nel mondo di oggi, né, a maggior ragione, è possibile subordinare la tutela dei diritti umani alle esigenze dei rapporti economici e industriali. Le due cose si tengono insieme. Il rafforzamento della democrazia e delle libertà fondamentali, la tutela della persona e dei suoi diritti inalienabili sono valori che qualificano la civiltà, 1'affidabilità e il grado di sicurezza di un Paese e ne garantiscono lo *status* di *partner* industriale e commerciale serio e credibile, cosa che non avviene in caso contrario. Viceversa, i programmi più virtuosi ed efficaci di collaborazione e cooperazione economica, sociale e culturale aiutano il consolidarsi di un nuovo clima democratico e civile in queste società e danno speranze ai giovani, alle donne, alla società civile. L'Egitto - lo ribadiamo L'Egitto - lo ribadiamo - è un Paese cruciale in un'area terribilmente complessa e delicata. I nodi della Libia, di Israele e Palestina, della Siria sono lì a ricordarcelo. Ma un ruolo di potenza regionale equilibrante e attiva contro il fondamentalismo si svolge appieno se si dimostra di operare perché la democrazia, la giustizia, i diritti umani essenziali siano garantiti e facciano parte di un patrimonio culturale e istituzionale solido e sicuro. Il Governo assuma, dunque, tutte le iniziative necessarie, sviluppi ogni forma di pressione morale, diplomatica ed istituzionale. Valuti l'Esecutivo i passi giusti da fare, ma nessuna misura politica e relazionale sia esclusa pur di raggiungere l'obiettivo.

della magistratura di Potenza svela l'operato di un comitato d'affari, garante degli interessi di compagnie petrolifere, in special modo della Total, come si evince dalle intercettazioni di società legate al compagno dell'ex ministro Guidi. L'emendamento, che è stato inserito nella legge di stabilità e poi riportato nel maxiemendamento presentato...

proprio il Movimento 5 Stelle ha denunciato, in quest'Aula, il 18 dicembre 2014, attraverso un intervento del senatore

con la Total. Questa Assemblea forse non si è voluto accorgere di quello che stava avvenendo. Proprio in merito a questo il Movimento 5 Stelle, dato il coinvolgimento dell'ex ministro Guidi, dell'onorevole Boschi (citata nelle intercettazioni, in cui si dice che vi è un accordo a livello governativo), dei vari sottosegretari del Governo (cito, oltre al ministro dello sviluppo economico Guidi, il sottosegretario *pro tempore* allo sviluppo economico, Simona Vicari e il sottosegretario di Stato alla salute, De Filippo) e del capo di stato maggiore della Marina militare, ammiraglio Giuseppe De Giorgi. Queste sono tutte le persone coinvolte nell'inchiesta: devono dare spiegazioni ai cittadini italiani e a questa Assemblea e, soprattutto, tutte persone che fanno parte di questo Governo. Quindi, il Movimento 5 Stelle chiede - non domani,

degli atti gravissimi che coinvolgono Governo, maggioranza e anche gli enti locali gestiti dal PD. Ricordiamo, infatti, a quest'Aula che è stato arrestato arrestato un ex sindaco del PD nel corso dell'indagine. Il Movimento 5 Stelle, per tutti questi fatti, e per la chiara responsabilità che ha il Governo, e anche la maggioranza (che ha consentito che quell'emendamento entrasse nella legge di stabilità malgrado le denunce del Movimento 5 Stelle), chiede che venga convocata immediatamente una Conferenza dei Capigruppo, nel dovuto rispetto

per andare in televisione e cercare di giustificare davanti al Paese quanto è moralmente ingiustificabile in qualsiasi altro Paese che possa dirsi democratico: ovvero, che ci sia un comitato d'affari al Governo del Paese. Un comitato d'affari presieduto da una persona non eletta! Questo è quanto sta accadendo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Noi avremmo voluto vedere qui oggi il presidente Renzi a rispondere delle accuse che la magistratura sta muovendo al suo Governo e delle posizioni torbide del ministro Boschi. Ricordo a lei, signora Presidente, che era presente come noi quella notte, che, quando fu votato il bilancio dello Stato e quando fu votata la finanziaria, tenne un Consiglio dei ministri proprio qui. Un Consiglio dei ministri alla presenza della ministra Boschi e della ministra Giannini, di modificare la Nota di variazione. Ancora una volta qui, in questo Senato, quali atti sono stati compiuti? La domanda vera è se sono stati compiuti reati. Noi vogliamo ci sia chiarezza, ma abbiamo già una chiarezza: il Governo del Paese merita ben altro spessore.

Perché qui si deve rispondere davanti ai cittadini e non davanti al proprio direttorio, che viene puntualmente umiliato. Si convochi una Conferenza dei Capigruppo e si metta subito all'ordine del giorno la discussione di una mozione di sfiducia di fronte alla quale il Governo deve rispondere.

come Sinistra italiana, abbiamo scritto al Presidente del Senato, perché trovavamo assolutamente necessario inserire immediatamente nel calendario del nostri lavori un dibattito. E chiedevamo appunto al presidente Renzi di venire immediatamente in Aula. Signora Presidente, non è possibile pensare che quest'Aula non possa avere una discussione nel merito di quanto accaduto e pensare di chiudere tutta la vicenda con le dimissioni del ministro Guidi. Il quadro che è emerso, e che sta continuando ad emergere, è il quadro molto preoccupante di una commistione tra interessi privati rivendicati quasi come interesse generale. Noi stiamo depositando anche la richiesta di una Commissione d'inchiesta parlamentare sulla vicenda, perché è evidente a tutti che il conflitto di interessi è enorme e che questo Governo e questa maggioranza non hanno mai voluto intervenire con una legge seria sul conflitto di interessi. Quando era all'opposizione, anche Renzi ha più volte accusato, anche il suo stesso partito, di non avere perseguito l'obiettivo di una legge seria sul conflitto di interessi, ma adesso questo elemento è completamente scomparso. È sotto gli occhi di tutti che la questione è enorme e merita non solo una discussione, ma anche di essere approfondita. Tanto più che le cose sono avvenute durante un procedimento legislativo all'interno del Senato, durante la legge di stabilità, dopo che alla Camera nello sblocca Italia

sia importante che anche in quest'Aula si possa dibattere degli accadimenti che hanno portato alle dimissioni del ministro Guidi. La mozione di sfiducia è uno strumento tipicamente parlamentare per far sì che questo possa avvenire

Signora Presidente, era inevitabile che all'apertura dei lavori dell'Assemblea questa settimana il tema prevalente dal punto di vista politico potesse essere questo. Quindi io, con la stessa serietà che ha distinto i colleghi che hanno richiamato l'obbligo di rispondere al Parlamento e l'obbligo che il Parlamento ha di occuparsi delle vicende più importanti, oltre che di quelle

quando c'è stata una richiesta d'arresto per un'attività che il collega aveva svolto come Presidente di Commissione. La magistratura opinava che alcuni comportamenti sui quali il Parlamento si era espresso fossero penalmente perseguibili; mi sembrava una cosa - anche se i colleghi del PD in Commissione avevano votato per l'arresto

per rimodulare o rifare la nostra flotta questo sarebbe un traffico di influenze illecite. Leggo poi che il ministro Pinotti sarebbe coinvolta nella vicenda perché, essendo eletta in Liguria, ed essendoci in Liguria La Spezia dove si trova parte della flotta, ecco che scatterebbe il reato. Avviso i colleghi di maggioranza e di opposizione che noi abbiamo subito come centrodestra infami iniziative delle procure tese a delegittimare la politica. Adesso, come capita agli apprendisti stregoni, quelli che hanno voluto norme folli come il traffico di influenze illecite incominciano a capire che cosa vuole dire quando si alzano polveroni incredibili.

ad un'autorizzazione a procedere per l'estrazione del petrolio o alle piattaforme in mare ed essere contrari a fatti di malcostume, che però vanno documentati per capire se c'è corruzione, se c'è concussione, se ci sono tangenti. Non si può teorizzare, come è stato fatto qui - e per questa ragione chiedo anch'io che i Capigruppo ci consentano

Signora Presidente, intervengo per esprimere apprezzamento per l'intervento del senatore Giovanardi: un intervento equilibrato di un parlamentare che, a prescindere che sieda nei banchi della maggioranza o dell'opposizione, esprime coerentemente il suo pensiero. Comprendo perfettamente la posizione del Movimento 5 Stelle, così come comprendo la posizione di altre forze, come SEL, però non riesco a capire la posizione di forze politiche che per anni, in questo ultimo ventennio, hanno gridato la necessità di avere una magistratura indipendente e una classe politica che potesse svolgere serenamente il proprio lavoro, senza subire attacchi attacchi molto spesso anche strumentali da parte della magistratura stessa. Ho sentito il collega della Lega Nord parlare di un procedimento che vedrebbe coinvolto il ministro Guidi come indagata. Non mi risulta questa notizia. Attenzione, colleghi, una volta il grande senatore Mancuso nell'Aula del Parlamento che la giustizia di popolo è giustizia tribale. Facciamo fare il lavoro a chi ne ha legittimità, facciamo lavorare la magistratura. Noi, certo, possiamo anche commentare l'episodio: sicuramente è stata inopportuna sicuramente è criticabile ed anch'io non ho alcuna difficoltà a criticare, sotto il profilo della correttezza istituzionale,

che con noi ha governato il Paese per molti anni ed ha gridato questa stessa esigenza di vedere la classe politica non destinataria di attacchi

Non voglio apparire persecutoria nei confronti del Gruppo Movimento 5 Stelle però, siamo in una situazione in cui un senatore per Gruppo, ad inizio di seduta e non nel corso della discussione, quando ciascun senatore può intervenire sull'ordine dei lavori, è intervenuto per chiedere la convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Su questo non si apre un dibattito. Le chiederei quindi, cortesemente, di rinunciare al suo intervento per non aprire un dibattito su questa vicenda, perché se lei interviene su quello che hanno detto gli altri, altri vorranno intervenire su quello che avrà detto lei e si apre un dibattito Le richieste dei colleghi, come ho fatto presente, saranno tutte immediatamente rappresentate al Presidente del Senato perché adotti le proprie determinazioni appena possibile. Quando passeremo all'ordine del giorno, che reca la discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto-legge ...

Grazie, signora Presidente. Intervengo sull'ordine dei lavori e secondo quanto previsto dall'articolo 92 del vigente Regolamento del Senato. Anche precedentemente poteva darmi la parola, perché il Regolamento così prevede.

non è un privilegio, è un diritto. Mi consenta di poter esprimere brevemente quanto volevo dire. Rispetto a quanto detto - e con questo non voglio aprire un dibattito, ma se il Senato vorrà farlo saremo ben lieti di che oltre alle persone che sono state e sono indagate per questa vicenda, risulta essere indagato - ed è altrettanto grave - anche il capo di stato maggiore della Marina, l'ammiraglio De Giorgi, che ha capi di imputazione molto gravi. Ne leggo solo alcuni: alcuni: associazione a delinquere, traffico di influenze e abuso d'ufficio. In questa situazione ricade anche la cosiddetta legge navale che ha stanziato ben 5,4 miliardi di euro per il rifacimento di navi e proprio questo provvedimento

Signora Presidente, io volevo intervenire proprio per sollecitare la Presidenza a passare all'ordine del giorno perché non è accettabile che i rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari, basandosi su notizie frammentarie e incerte anche dal punto di vista del contenuto giudiziario, trasformino quest'Aula in un tribunale. I tribunali sono da un'altra parte.

*relatore*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, questo importante provvedimento di riforma, che peraltro è stato oggetto di particolare attenzione (e colgo l'occasione per ringraziare il presidente Marino che, insieme alla Commissione finanze della Camera, ha promosso un seminario istituzionale per confrontarsi e discutere il progetto di autoriforma presentato dalla banche di credito cooperativo), ha suscitato e suscita attenzione e giudizi anche contrastanti, ma tuttavia deve essere inquadrato...

in un nuovo contesto rispetto al quale la funzione importante del sistema delle banche di credito cooperativo può essere preservata se abbiamo il coraggio di cambiare se invece ci attestiamo su una posizione di blocco o di resistenza ai cambiamenti perché in tal modo arrecheremmo un danno alla funzione vitale per la nostra economia reale

il contesto è completamente mutato, insieme alla lunga crisi che abbiamo attraversato e da cui abbiamo cominciato da poco ad uscire. L'unione bancaria è una realtà e con questa bisogna fare i conti. È una realtà perché c'è un apparato normativo importante, che ha un impatto forte su tutto il sistema bancario: il meccanismo di vigilanza unico, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, il meccanismo di garanzia dei depositi. Si tratta di un apparato normativo imponente, una volta messo sul mercato, ne ha modificato la natura, perché ha creato le condizioni per intervenire su una fragilità di sistema del nostro sistema bancario, che si è evidenziata durante questi lunghi anni di crisi. L'impatto normativo su questa particolare tipologia di banche, cioè le banche di credito cooperativo, è stato enorme e molto forte. La scelta, da parte dell'Unione europea, di un sistema di norme unico, comune ed omogeneo per tutti i tipi di banche naturalmente pone una serie di problemi, che non possono essere risolti solamente con adattamenti posteriori.

lo *SME supporting factor*, un risultato importante per il nostro Paese, che ha consentito e consente di avere un assorbimento di capitale delle banche meno oneroso, a fronte di finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese. Questo è un elemento che va conservato ed ampliato; gli effetti sono stati valutati molto positivamente dal sistema delle banche di credito cooperativo. Tale valutazione verrà rinnovata in sede europea, con la relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio

di trovarsi di fronte a meccanismi più stringenti sul tema dell'erogazione del credito, crea altri elementi

tempo, di svolgere con strumenti nuovi le funzioni che è chiamato ad assolvere. Tali funzioni impongono necessariamente, come tutte le altre articolazioni del sistema bancario, una patrimonializzazione più forte e quindi una garanzia di fronte al rischio della problematica connessa

pari a quasi il 56 per cento del totale delle banche operanti in Italia, con 4.414 sportelli, 1.248.000 soci. Sono presenti in 101 Province, in 2.693 Comuni; in 549 Comuni sono l'unica presenza bancaria. Hanno 31.000 dipendenti. Nel 2015, su 130 miliardi di euro di finanziamento alla clientela, 85 sono stati erogati alle imprese. Nel periodo di crisi, dal 2010 al 2015, i finanziamenti erogati dalle banche di credito quindi, una caratterizzazione in senso positivo, a fronte, invece, di una riduzione di circa 56 miliardi del resto dell'industria bancaria. La lunga recessione che ha colpito il sistema produttivo ha naturalmente peggiorato la qualità del credito. La raccolta della clientela ha superato i 161 miliardi e il patrimonio delle banche di credito questo sistema presenta delle criticità, anche superiori alla media, per alcuni aspetti. La redditività del sistema delle banche di credito cooperativo, proprio per la tipologia di clientela che viene servita, ha risentito moltissimo della lunga crisi dell'economia reale. I bassi tassi d'interesse, la domanda stagnante, il crescere del volume delle partite deteriorate hanno compresso i margini di intermediazione e la stessa difesa dell'occupazione (abbiamo parlato di 31.000 dipendenti) naturalmente ha reso rigidi i costi.

L'azione riformatrice del Governo - voglio ricordarlo - è andata proprio nella direzione di un rafforzamento nei fondamentali del sistema, con una serie di riforme: la riforma delle banche popolari, l'autoriforma delle fondazioni, il rafforzamento del sistema finanziario, la garanzia pubblica sulle *tranche senior* di cartolarizzazione dei crediti non performanti. L'obiettivo, quindi, è sostenere l'economia reale sfruttando la politica espansiva della BCE. Infatti, la contraddizione risiede proprio a fronte di una enorme massa di liquidità disponibile grazie alla politica espansiva della BCE, le regole più stringenti di accesso al credito e di patrimonializzazione delle banche restringono la possibilità

sia attraverso il passaggio del decreto-legge, sia attraverso le modifiche apportate in sede di conversione, si sono colti gli obiettivi fondamentali della riforma. un decreto-legge che già recepiva le indicazioni del progetto di autoriforma, in particolare sulla *governance* del capitale della banca capogruppo e su altri aspetti importanti. A fronte dell'*iter* parlamentare di conversione con le modificazioni, vi sono tutta una serie di elementi che possiamo sottolineare, insieme agli aspetti salienti già contenuti nel decreto. Intanto, l'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo viene consentita solo attraverso imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Questo è il primo elemento. È conservato e rafforzato il carattere della mutualità: non viene meno. Anzi, sono ribaditi tutti i connotati della mutualità delle banche di credito cooperativo: l'operatività, la prevalenza, il rapporto con i soci, la destinazione degli utili e la disciplina fiscale.

Il controllo della capogruppo è in mano alle banche di credito cooperativo che detengono in misura maggioritaria il capitale. C'è la graduazione dei poteri della capogruppo in relazione alla meritevolezza delle singole banche di credito cooperativo, al fine di ribadire la connessione con le finalità mutualistiche dei poteri della capogruppo, i quali sono proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti. Il requisito minimo del patrimonio della capogruppo, per dare unità e solidità al sistema, è stabilito in un miliardo di euro. Dobbiamo tener conto che l'indicazione di un miliardo di euro cerca di dare risposta a due elementi.

alle nuove necessità del mercato e al nuovo apparato normativo che ho prima citato. Nello stesso tempo, a fronte di una platea di banche di credito cooperativo che hanno un patrimonio complessivo di 20 miliardi di euro, non si è voluto escludere che si possano realizzare più gruppi. C'è un protagonismo delle banche di credito cooperativo con l'attribuzione all'assemblea dei soci delle singole banche del potere di nominare i propri organi sociali. È consentita la costituzione in gruppi bancari cooperativi nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Altra novità è la possibilità di creare sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni all'interno del gruppo bancario cooperativo. La soglia di un miliardo di euro di patrimonio, che ho prima ricordato, è quindi prevista per favorire un'aggregazione amplia, ma non esclusiva. La soglia dei 200 milioni di euro di patrimonio per approfittare del meccanico della *way out*

Le banche che hanno questo requisito a livello patrimoniale sono 14 e interessano diverse aree del Paese.

in realtà si mette ordine nel sistema e si fa chiarezza. Un elemento molto importante riguarda l'estensione della garanzia pubblica sulla cartolarizzazione delle sofferenze anche agli intermediari finanziari. previste regole più flessibili per utilizzare gli sconti fiscali nell'acquisto di una casa messa all'asta. Un altro elemento importante, che avevo tralasciato e che invece voglio sottolineare, il quale era anche stato sollecitato dal sistema delle banche di credito cooperativo rispetto alla previsione contenuta nel decreto‑legge in esame, attiene al fondo temporaneo a sostegno dell'attività di credito cooperativo, che, in attesa della costituzione di un nuovo gruppo, può intervenire come strumento mutualistico-assicurativo per consolidare il sistema delle Il termine di sessanta giorni per chi vuole avvalersi del meccanismo della *way out* implica che l'affrancamento delle riserve senza devoluzione del patrimonio deve essere evento evento che non può essere improvvisato e che può essere utilizzato solo da soggetti strutturati per poterlo fare. In questo ambito il ruolo di vigilanza della Banca d'Italia è molto importante. La Banca d'Italia ha un ruolo molto forte e pregnante perché definisce i requisiti minimi organizzativi della capogruppo e il contenuto minimo dei contratti di coesione. Il MEF prevede con decreto una soglia minima di partecipazione alla capogruppo

per rimanere competitivo sul mercato, per tutelare i cittadini, le imprese e i loro risparmi. Se noi rinunciassimo alla volontà di riforma e di innovazione del sistema,

che serve a fare chiarezza rispetto a una norma approvata alla Camera e che riguarda l'aspetto degli assegni bancari. L'articolo 17-*ter* del presente provvedimento, come modificato alla Camera,

per gli assegni presentati in forma elettronica, di produrre per il protesto una dichiarazione sostitutiva della Banca d'Italia, richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti come alternativa al ricorso al notaio.

complessivamente volte a consentirne la circolazione e il pagamento anche in forma elettronica. In particolare, il numero 2 della citata lettera *b)* dispone che il rifiuto del pagamento possa essere constatato oltre che con atto autentico (protesto o dichiarazione del trattario dell'assegno bancario) anche con dichiarazione della Banca d'Italia in qualità di gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, la quale attesti che l'assegno bancario presentato in forma elettronica non è stato pagato. La lettera *c)* del citato comma 7 stabilisce l'equivalenza, a ogni effetto di legge, delle copie informatiche degli assegni cartacei rispetto agli originali da cui sono tratte, a condizione che la loro conformità all'originale sia assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche stabilite con decreto ministeriale. Alla Banca d'Italia è demandato il compito di emanare, entro dodici mesi dal predetto decreto, apposito regolamento per la disciplina delle regole tecniche e per l'applicazione delle disposizioni in esame del decreto ministeriale. Ai sensi della lettera *f)* del citato comma 7, il complesso delle modifiche sopra descritte entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del predetto regolamento della Banca d'Italia. La citata disciplina farebbe esplicito riferimento ai soli assegni presentati in forma elettronica e non anche agli assegni cartacei per i quali si stabilisce l'equivalenza, ad ogni effetto di legge, delle copie informatiche rispetto agli originali da cui sono tratte, a condizione che la conformità all'originale sia assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria forma digitale. Il regolamento della Banca d'Italia per la disciplina delle Il regolamento della Banca d'Italia per la disciplina delle regole tecniche non è stato emanato entro il termine previsto dal decreto-legge n. 70 del 2011 e la possibile emanazione successiva all'entrata in vigore dell'articolo 17-*ter* del provvedimento in esame comporterebbe la reintroduzione della normativa che lo stesso articolo 17-*ter* intende superare, producendo così un'implicita abrogazione per il principio della legge posteriore. Peraltro, il consenso alla corretta interpretazione della norma conforme dell'articolo 17-*ter* del provvedimento in discussione si è manifestato anche in sede d'esame al Senato del disegno di legge sulla concorrenza con l'approvazione dell'emendamento che interviene modificando il citato articolo 8, comma 7, lettera *b)*, numero 2 del decreto-legge n. 70, convertito con modificazioni, nella legge n. 106 del 2011 e replicando quanto previsto dal citato articolo 17-*ter* al fine di prevederne l'entrata in vigore con la pubblicazione del regolamento della Banca d'Italia; ed evita in tal modo che la suddetta pubblicazione del regolamento riporti in vita una normativa superata.

piuttosto complicata da ricondurre ad equità ed è un dato che fornisce il senso e il merito

rappresenta uno stigma, una ferita fortissima per l'attività legislativa di questo Governo. Lo voglio dire non a caso, signora Presidente e colleghi: anche quando i contenuti hanno un senso, se il contenitore non ce l'ha o è palesemente illegittimo è impossibile dare un senso di legittimità ai contenuti stessi. Ancora una volta ringrazio il collega Moscardelli per aver tentato di spiegare come il Governo vuole risolvere il problema delle banche di credito cooperativo, cooperativo, che peraltro non definirei di bruciante attualità, esattamente come non abbiamo definito di bruciante attualità il tema delle banche popolari. di questo anno bancario, vissuto molto pericolosamente dal Governo Renzi, è purtroppo una modalità autoritaria e dirigistica di imporre al sistema bancario delle regole assolute, che valgono - ahimè - soprattutto per alcuni territori, su cui il Presidente del Consiglio e alcuni Ministri "di peso" del suo Governo amano molto operare. Vi assicuro, signora Presidente e colleghi, che né nell'illustrazione di questa questione pregiudiziale, né nel prosieguo della discussione lasceremo cadere questo riferimento, senza darvi un'opportuna motivazione.

quando si fanno riforme organiche e di sistema, annunciate da venti anni, tentate e inserite in cassetti polverosi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per poi essere ritirate fuori e proditoriamente inserite nel veicolo del decreto-legge. Abbiamo detto più volte che questo viola in maniera palese, marchiana e intollerabile, per quanto ci riguarda, le caratteristiche costituzionali previste in maniera implacabile e ineludibile dall'articolo 77, che non può essere modificato per via convenzionale o perché al *Premier* piace il decreto-legge. Colleghi, con tutto il rispetto del mondo per l'inquilino del Colle e per ciò che avviene sul Colle più alto, è francamente imbarazzante pensare che tutto questo sia controfirmato da chi ha ha posto come cifra del suo mandato il fatto di limitare l'uso improprio della decretazione d'urgenza o l'uso del decreto-legge sulla base di una generica, inesistente urgenza nel provvedere. Basta leggere il titolo di questo provvedimento, perché ormai i titoli stessi

disorganiche, estremamente indigeste per queste Camere e assolutamente indigeribili, tossiche e anche un po' velenose, che vengono proposte da parte di chi ritiene forse di esercitare, più che una *premiership*, un ruolo di autoritativa organizzazione del contenuto dei provvedimenti. Mi spiego meglio. Anche Anche per quanto riguarda questo decreto-legge in materia bancaria, ricordo che tutti i decreti-legge in materia bancaria che hanno attraversato queste Aule sono stati caratterizzati, oltre che dall'uso di uno strumento improprio e assolutamente incostituzionale, anche dall'uso della fiducia, altro strumento ugualmente improprio e incostituzionale nell'ottica di una riforma di sistema e di un rapporto che avrebbe dovuto essere molto più intenso, fiduciario, collaborativo e cooperante con tutti noi parlamentari.

fa, che mai una riforma organica e di sistema può essere attuata con un decreto-legge. Colleghi, guardandoci negli occhi e mettendoci una mano sulla coscienza, non abbiamo bisogno che ce le dica la Corte costituzionale. Sappiamo tutti benissimo che, per modificare un testo unico, qual è quello in materia bancaria, non servono i decreti-legge ma disegni di legge ugualmente omogenei, strutturati, coordinati e condivisi, che diano la misura di una riforma che non si attua mai, se organica e strutturale, in maniera simultanea, ma attraverso stadi, provvedimenti e procedimenti attuativi successivi.

ho apprezzato molto il tentativo, quasi da zingara con la palla di cristallo, di preconizzare i modelli di *governance* che caratterizzeranno questa *holding* del sistema di credito cooperativo. Ma come facciamo a sapere ciò che non è ancora scritto,

con l'uso del decreto-legge. Come incompatibile con l'uso del decreto-legge è l'utilizzo addirittura di atti di natura non regolamentare, che non piacciono né alla Corte costituzionale né al Consiglio di Stato e che, invece, al legislatore piacciono da morire, tanto che ne fa un uso quasi sconsiderato.

L'Europa non ci chiede di fare dei conglomerati capigruppo aspirapolvere che riportino nel loro grembo tutte le tutte le banche di credito cooperativo sulla base di una valutazione non per merito, non per aggregazione territoriale, provinciale, di specifiche di erogazione del credito di prossimità, ma solo per valore. Elemento che, peraltro, violerebbe una serie di principi costituzionali quali: l'articolo 3, il principio di uguaglianza; l'articolo 45, il principio mutualistico, che noi tutti sappiamo dover essere senza scopo di lucro, senza fini speculativi, caratterizzato dalla sua natura e dai suoi fini sociali, pervertiti da questo schema. Cito poi l'articolo 47 sulla tutela del risparmio, e l'articolo 53 sulla progressività della tassazione, che viene meno sulla base dell'imposizione di una

per fare una considerazione di merito che ci riserviamo di estrinsecare e spiegare molto meglio nell'ambito della discussione generale, che sarà - ahimè - molto breve, perché purtroppo il treno della riforma come sempre passerà oltre la stazione Senato, e noi potremo dare solo la fiducia, non discutere nel merito e non cambiare niente: è una caratteristica costante ormai della nostra attività. Però, signora Presidente, colleghi, per quale motivo ancora una volta andiamo controtendenza rispetto ai Paesi che funzionano in Europa? La Francia, la Germania, l'Olanda, ma anche il Canada (dando a questa considerazione una dimensione extraeuropea), tengono tengono da conto le loro banche di credito cooperativo come erogatrici di crediti di prossimità che consentono di tutelare l'economia reale e di contrastare gli *shock* economici. Colleghi, ancora una volta stiamo andando in controtendenza, nostro malgrado, perché noi non aderiamo a questa iniziativa legislativa: non siamo stati sufficientemente consultati, non ci piace il metodo e non ci piace il merito, e andiamo verso una deriva non condivisa e non condivisibile, in controtendenza rispetto a un'Europa che non possiamo usare solo quando quando ci fa comodo. Per tutti questi motivi chiediamo che non si prosegua ulteriormente nell'esame di questo provvedimento.

o a fare finta di idolatrare la Costituzione; noi vogliamo parlare seriamente di un problema che sta affliggendo questa legislatura.

Dobbiamo comunque ricordare, se vogliamo essere dei legislatori e non qualcosa di diverso, che l'articolo 70 della Costituzione affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere. Ciò che invece continuiamo a vedere e a cui stiamo andando incontro è un vero e proprio svuotamento e una mortificazione delle attività del Parlamento, con una concreta impossibilità, anche da parte dell'opposizione, di partecipazione a un confronto e a un dibattito politico, e di esercitare la propria funzione, che è quella del controllo politico. Non dovete pensare che l'opposizione dia solo fastidio; l'opposizione è nata per esercitare un controllo. E da questo dibattito non riusciamo a rendere effettiva la democrazia.

l'abbiamo visto anche e soprattutto sui provvedimenti che riguardavano la giustizia, di cui non si comprende nemmeno quale potesse essere il requisito di necessità e urgenza, visto che i problemi della giustizia affliggono i tribunali da molti anni. Ricordiamo che, in realtà, i disegni di legge di iniziativa parlamentare arrivano a un approdo positivo solo nell'1 per cento

doveva mettere in pratica quelle norme, eseguire quello che veniva detto dal Parlamento. Sta succedendo esattamente il contrario: è il Governo che dice cosa deve fare il Parlamento.

ci si chiede quale possa essere la necessità e l'urgenza di intervenire su un sistema come quello bancario, con particolare riferimento a ciò che stiamo esaminando in questo decreto-legge. Ci si domanda il perché di questa famosa urgenza. Ricordiamo che probabilmente sono tra 15 e 17 le banche che potrebbero avere elementi patrimoniali di criticità fatali, e che questa fatalità potrebbe esercitarsi nei prossimi diciotto mesi, su un totale di

parla di esclusione dalla tassazione dei contributi percepiti dai soggetti per cui risultino attivate procedure concorsuali, nonché, in un altro Capo, si modifica il testo unico sulla intermediazione finanziaria. Stiamo parlando di tematiche

soprattutto quando vediamo che con alcune disposizioni si prevede che la banca di credito cooperativo che viene esclusa dal gruppo bancario possa continuare la propria attività solo mediante una sua trasformazione in società per azioni.

chiediamo che non si proceda all'esame del disegno di legge in ci troviamo per l'ennesima volta ad illustrare una pregiudiziale di costituzionalità per un provvedimento che riguarda le banche. Banche e petrolio, oro verde delle banconote e oro nero del petrolio, sono i due interessi principali di questo Governo. Brucia ancora la ricapitalizzazione di Bankitalia, avvenuta con un vero e proprio *blitz* alla Camera dei deputati e che ha visto un regalo di oltre 7 miliardi di euro alle banche. Ed è ancora in ballo il decreto legislativo che permetterebbe alle banche di appropriarsi della casa di chi non riesce a pagare qualche rata, senza passare dal vaglio di un giudice. E mentre su Monte dei Paschi di Siena ancora non si fa luce, ecco la truffa delle banche di credito cooperativo. Mentre tutti si aspettavano un provvedimento per salvaguardare i risparmiatori truffati, ecco un provvedimento che, da una parte, ecco un provvedimento che, da una parte, mette in sicurezza le banche e, dall'altra, per colpa di qualche farabutto, punisce il sistema del credito cooperativo, l'unico che manteneva ancora alta la sua funzione di emissione di credito. Era il 19 febbraio 2014 quando Beppe Grillo, seduto al tavolo con Renzi, gli disse, senza usare mezze parole: «Tu rappresenti le banche». Mai parole furono più azzeccate e profetiche. Questo Governo è il Governo delle banche e dei banchieri, è il Governo della famiglia Boschi, della massoneria toscana e non solo. È il Governo delle *lobby* del petrolio, delle *lobby* delle assicurazioni, dei grandi produttori di energia, è il Governo dei conflitti di interesse. Con Berlusconi pensavamo di aver toccato il fondo, ma Renzi ha scavato di più, sempre di più. Il decreto-legge che oggi chiediamo di non esaminare presenta profili di incostituzionalità. Vorrei solo ricordarvi che la sentenza n. 220 del 2013 della Corte costituzionale del 2013 - non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, concepiti dal legislatore per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall'insorgere di «casi straordinari di necessità la trasformazione per decreto-legge dell'intera disciplina ordinamentale appare incompatibile, sul piano logico e giuridico,

Ma qualcuno ci ha visto il caso straordinario di necessità e di urgenza. Peccato che poi alcune norme, la banca che intende assumere il ruolo di società capogruppo dovrà sottoporre alla Banca d'Italia

discuterne serenamente, ognuno con le proprie opinioni, invece, come accade ormai di solito,

tanto votano qualsiasi cosa, quindi potremmo evitare anche di fare le riunioni di questo decreto‑legge è in contrasto con gli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione.

Perché non predisponiamo alcune norme, come vi stavo dicendo prima, che tutelino il risparmio, che vietino la vendita di prodotti finanziari deteriorati a

un'interpretazione autentica di come si dovevano trattare i patrimoni delle cooperative che si scioglievano o che si trasformavano: il patrimonio doveva andare ai fondi statali. Invece noi che facciamo? Diamo loro l'opportunità di tenersi il patrimonio e di versarne solo una parte, ossia il 20 per Mi chiedo peraltro con quale titolo venga chiesto questo 20 per cento del patrimonio netto. Cos'è? Una penale, una tassa, un contributo? Qualcuno ce lo spiegherà, a noi o alla magistratura, mi auguro. Con questo trucchetto si va anche ad interferire sul diritto alla concorrenza, perché le cooperative che vengono sciolte e si trasformano vengono ancora assoggettate all'interpretazione autentica, mentre le BCC no. Quindi c'è una piccolissima

Dobbiamo attendere che l'Europa ci dica qualcosa, o ci risponde il Ministro, per tranquillizzarci? PRESIDENTE.

ancora una volta che in questo Paese non esiste più la democrazia e non esiste più il Parlamento, che non serve a nulla ed è un mero esecutore degli ordini del Governo. Questo è avvenuto e continua ad avvenire da anni, nella vostra più totale indifferenza. Dante la chiamava "ignavia" e metteva gli ignavi nel girone più duro, con la pena più dura, perché considerava l'ignavia il peggiore dei peccati. La storia non dimenticherà questa stagione e non dimenticherà voi, ignavi in alcuni casi, complici e collusi in altri casi. Abbiate un ultimo sussulto di coraggio, provate ad alzare la testa da quel banco e leggete cosa state votando. Non fate come con la legge di stabilità 2015, che avete votato nonostante ne mancasse un pezzo, per non parlare poi del cosiddetto emendamento Total-Total. Provate a capire e non fatevi distrarre distrarre dalle sirene delle banche, perché al massimo per voi arriveranno le sirene della polizia. Salutiamo gli allievi e i docenti dell'Istituto comprensivo «Mazzini-Capograssi» di Sulmona, in provincia dell'Aquila, che sono in visita al Senato. Benvenuti.

noi siamo qui, ancora una volta, nella distrazione più totale dell'Assemblea, a porre una questione pregiudiziale su questo disegno di legge di conversione dell'ennesimo decreto-legge. Quello che francamente, signora Presidente, deve continuare a

evidentemente conversando di banche o di Basilicata e noi continuiamo a intervenire su questioni che non sono di poco conto, come di questo disegno di legge di conversione dell'ennesimo decreto‑legge, che impatterà sul futuro del nostro Paese, sull'economia e sugli interessi di tanti risparmiatori. Peraltro, tutto l'*iter* di questa riforma delle banche di credito cooperativo e disposizioni relative alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (per non parlare ovviamente del regime fiscale relativo alle procedure di crisi,

il Parlamento che avrebbe dovuto, poi, assumere delle decisioni. Vi sono state, peraltro, interrogazioni e richieste ai Ministri competenti di venire a riferire, ma questo non è accaduto. è accaduto. Questa discussione e le varie proposte di autoriforma che erano state avanzate sono la prova provata che evidentemente non era possibile utilizzare il decreto‑legge.

ed è dedicato soltanto ad intervenire in modo necessitato e urgente per dare risposte rapide a situazioni che debbono essere fronteggiate immediatamente. Per questo motivo il legislatore ordinario, con una norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere misure di immediata applicazione.

una riforma di sistema, quindi non un intervento di necessità e urgenza e di immediata applicazione, ma una riforma complessiva e non di poco conto?

bancario e quindi posso capire che voglia utilizzare il decreto‑legge, ma è assolutamente improponibile. La Corte costituzionale, tra l'altro, con la sentenza n. 220 del 2013, che è tassativamente esclusa la possibilità di ricorrere al decreto-legge quando si tratta di realizzare una riforma organica, come quella che è contenuta Il provvedimento, nel merito, detta una disciplina per un universo di 364 banche, tra quelle di credito cooperativo e le casse rurali, che costituiscono (con i loro 4.403

in una situazione anche complessa, certamente di casi non tutti brillanti, ha lavorato all'interno di un tessuto di economia reale.

che applica alla cooperazione di credito l'obbligo di partecipare a un rigido patto di coesione a un gruppo bancario unico con poteri di indirizzo e controllo sulle partecipate, quale precondizione per vedersi confermata l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia a esercitare il credito come banca di credito cooperativo. Questo vale a meno che non si dimostri di avere risorse patrimoniali superiori a 200 milioni di euro e di poter versare un'imposta straordinaria pari al 20 per cento, pena la liquidazione. È evidente, quindi, che da questo punto di vista c'è un obbligo che si configurerebbe, specie in assenza di una norma specifica che consenta la trasformazione in un altro tipo di banca senza devolvere le risorse patrimoniali, come una vera e palese violazione del dettato costituzionale, nonché

Vi è poi una questione molto seria, perché noi riteniamo che il principio di sussidiarietà nel settore del credito esca fortemente compromesso, posto che nel decreto‑legge in esame il trattamento di quelle banche

doveva essere addirittura rimesso in capo allo Stato stesso. In questo modo, con il semplice pagamento cento si verrà a creare un meccanismo chiaramente speculativo, che tradisce lo spirito dello statuto cooperativo e solidaristico. Per tutti questi motivi, crediamo

parte mira sostanzialmente a mettere in discussione un uso spregiudicato e indiscriminato, a detta di chi lo afferma, del decreto-legge; dopodiché si affrontano nel merito i temi dell'urgenza e della straordinaria necessità per poi entrare in modo scomposto anche sulle questioni di merito che, invece, saranno affrontate più precisamente nella discussione generale. È vero, l'Italia, rispetto a tanti

come Partito Democratico, insieme a tutte le altre forze che con noi reggono la legislatura, attraverso le riforme costituzionali.

dell'utilizzo del decreto-legge per fare in modo che ci siano dei tempi certi nelle discussioni dei provvedimenti legislativi. Venendo al secondo punto, che è quello della sussistenza

delle nuove norme che cercano di affrontare il tema delle crisi bancarie. Il 1° gennaio è già passato e, quindi, siamo già nel regime previsto dalla direttiva europea. In particolare questa direttiva preclude

ragioni forti e palesi di interesse pubblico e cioè l'esigenza di preservare la stabilità del sistema finanziario. È evidente che ciò non accadrà più tanto facilmente e quindi si andrà sicuramente incontro a casi che verranno risolti con il dissesto. Occorre fare in fretta per modificare il nostro sistema, per facilitare l'accesso al mercato dei capitali. al mercato dei capitali. La BRRD mira ad evitare l'utilizzo di risorse pubbliche ingenti in favore di banche in difficoltà, introducendo il principio generale in base al quale i costi delle crisi dovranno essere sostenuti dagli azionisti e dai creditori delle

l'Italia non ha utilizzato fondi pubblici per aiutare le banche. Oggi dobbiamo andare a ristrutturare e a rafforzare il nostro sistema bancario, per dare maggiori garanzie e tutele ai risparmiatori. Il ruolo della Banca d'Italia è noto e si esplica tipicamente nell'intervento ai primi segnali di deterioramento delle condizioni finanziarie, con la nomina di commissari che affiancano o sostituiscono gli organi di amministrazione. In caso di dissesto ci sono le procedure di liquidazione coatta amministrativa, ma nascono con questa direttiva anche delle speciali procedure per ridurre i rischi sistemici, trasferimento forzoso di beni dall'intermediario in crisi ad acquirenti privati, la costituzione di società veicolo, come le *bridge bank* o - peggio - le *bad bank*, e vi sono strumenti nuovi di risoluzione. Il *bail in*, spesso citato, è la riduzione forzosa del valore delle azioni e la conversione di alcune tipologie di debiti in azioni. Esso è il contrario del *bail out*, cui i costi vengono assunti dallo Stato. Non vengono colpiti dal *bail in* i depositi inferiori a 100.000 euro e quindi ci sono misure che tutelano comunque i piccoli risparmiatori. questo contesto mutato a richiedere di intervenire con urgenza affinché il sistema bancario e i suoi sottosistemi rafforzino la tutela dei risparmiatori,

In conclusione, con il provvedimento in esame è stato fatto un buon lavoro, proprio al fine di aumentare le tutele per i risparmiatori, promuovendo l'aggregazione delle BCC in uno o pochi gruppi bancari ben capitalizzati e capaci di attrarre gli investitori.

interpretato nel suo rigore letterario, così come credo abbia fatto la senatrice De Petris, ma come fanno tutti coloro che presentano una pregiudiziale di costituzionalità. Come ha detto bene il collega che mi ha preceduto, il primo punto che viene evidenziato in una questione di pregiudizialità di pregiudizialità costituzionale di un provvedimento è la possibilità, per quella materia e per quella norma, di vedere applicato il sistema di decretazione d'urgenza previsto appunto dall'articolo 77. Ma nella storia e nella prassi parlamentare abbiamo visto come questa norma sia stata, da tutte le forze politiche che si sono avvicendate al Governo del Paese, interpretata nella maniera più più elastica possibile. Ciò non significa - attenzione - violazione della norma costituzionale. Significa interpretare la norma sulla base di principi di ragionevolezza e di coerenza. Ora, si tralascia di considerare che la stessa norma, quando prevede la possibilità, ovvero il potere, del Governo di emanare un decreto-legge, attribuisce al Governo, autore di questo

sotto la sua responsabilità». Quindi, quando un Governo adotta un decreto-legge, ritenendo che siano sussistenti quegli elementi di necessità e di urgenza, lo fa anche assumendosi la responsabilità della sua azione legislativa. Allora, vista in questa direzione e visti i precedenti, mi pare che questa prima eccezione di incostituzionalità possa essere tranquillamente archiviata e licenziata senza essere meritevole di ulteriore approfondimento. Rimane il problema di merito e dell'urgenza: se vi sia o meno l'urgenza. Qui c'è una questione di punti di vista. Che cosa significa che vi è l'urgenza di intervenire o non vi è l'urgenza d'intervenire? Probabilmente, per qualcuno che mi ha preceduto si dovrebbe intervenire in caso di urgenza quando si sia verificata la crisi del settore o siano stati compromessi gli interessi dei risparmiatori. che il nostro Paese è il Paese principe della cultura del risparmio e quindi l'azione di Governo va, in questo ambito, nella direzione primaria, principe, di tutela dei risparmiatori, perché rappresentano una gran parte degli italiani. Allora, se bisogna intervenire quando si è verificata la crisi, cioè quando il malato sta morendo, forse, così ragionando, hanno perfettamente ragione i colleghi che mi hanno preceduto. Ma se vi è la saggezza di un intervento nella fase prodromica alla crisi e quindi alla irreversibilità del danno, allora questo è quel momento. Se abbiamo la direttiva n. 59 del 2014 che entra in vigore dal 1° gennaio 2016, qualcuno mi deve dire se, nell'arco di questi sei mesi, questa nostra architettura costituzionale, sarebbe stata in grado di intervenire adeguando le norme nazionali alla suddetta direttiva. Io sfido chiunque a dirmi che ciò non sarebbe stato possibile. E allora che cosa rimane, se non vi è la possibilità di un intervento normativo ordinario? Vi è la possibilità dell'intervento urgente del decreto-legge, non perché sosteniamo il Governo, ma perché, provvedimento per provvedimento, noi impegniamo la nostra ragione e la nostra saggezza nel decidere se condividere o non condividere; e in questo caso le nostre ragioni e il nostro senso di equilibrio

pregiudiziali che sono state presentate. e tante tessere. Magari i colleghi sono alla *buvette*. In questo modo evitiamo polemiche. Prego inoltre di adempiere all'indicazione della Presidenza di portare con sé le tessere quando ci si allontana

Signora Presidente, ci troviamo di fronte per l'ennesima volta a un provvedimento sul quale il Senato non si può esprimere.

grande è bello, secondo questo Governo: bisogna accorpare tutto; bisogna accorpare Comuni e banche. Purtroppo però nei grandi Comuni come nelle grandi banche spesso non abbiamo grandi buoni esempi. Allora quando vediamo grandi banche come, ad esempio, il prestigiosissimo Monte dei Paschi di Siena, di dimensioni più che ragguardevoli, oltre che di storia lunghissima, essere nelle condizioni in cui è, direi che non è desiderabile che altre banche seguano questo esempio. al Governo piacciono le grandi dimensioni, così probabilmente la politica ci può entrare più facilmente, o meglio quella politica del Governo ci può entrare più facilmente. piace anche l'anatocismo (che, benché sia una parola piuttosto ricercata, comincia a essere conosciuta dagli italiani, in particolare dai risparmiatori) che è il cosiddetto interesse sugli interessi. C'era una norma che lo vietava. Ebbene, alla Camera, con un bell'emendamento, è stato introdotto invece un comma, che oggi costituisce l'articolo 17*-bis* del provvedimento, che reintroduce l'anatocismo, sia pure solo su base annuale. Il bello è che, con notevole, straordinaria faccia tosta, viene presentato come una nuova abolizione, esattamente come nel comizio di Cetto La Qualunque, che promette l'abolizione della tassa sui cani e a chi gli fa presente che è già stata abolita risponde che l'abolirà di nuovo: abolita due volte! Ecco, peggio di Cetto La Qualunque, anziché abolire due volte, reintroduce ciò che era stato abolito, ovvero gli interessi sugli interessi: una norma di legge che c'era prima, reintrodotta a favore delle banche e contro il risparmiatore, specialmente il risparmiatore indebitato che può essere indebitato, nella maggiore parte dei casi, per produrre qualcosa, per comprare qualcosa; in altre parole, per far camminare l'economia. tra l'impresa, il commerciante, il professionista e la banca, il Governo si schiera apertamente dalla parte delle banche, raccontando di avere abolito l'anatocismo. Peccato che fosse già stato abolito e che in questo momento viene reintrodotto. (*Segue* MALAN). Il Senato non può intervenire perché in Commissione non è stato possibile fare alcun cambiamento; in Aula non si potrà intervenire perché io prevedo, con grandi capacità divinatorie, che, guarda caso, verrà posta la fiducia. In questi giorni si evidenzia come questo meccanismo della fiducia sia la totale cancellazione sia della trasparenza che dell'esame da parte del Parlamento. Il Governo vuole fare un favore alle banche? È libero di farlo, però deve poter affrontare

rischiando qualcosa da parte dei *leader* del proprio partito, potrebbero anche votare dalla parte dei cittadini e non necessariamente dalla parte delle banche. Tuttavia, questo non sarà possibile con il voto di fiducia, che ci viene giustificato con il fatto che bisogna fare in fretta. Ma qual è la fretta? Il decreto-legge

sono già in vigore. Ci sarebbe il tempo - visto che il decreto-legge scade il 15 aprile - di fare alcuni cambiamenti, per esempio, abolire sul serio l'anatocismo, e invece non lo si vuole fare: si pone la fiducia perché si deve fare in fretta. Abbiamo visto come si è fatto in fretta sul Tempa Rossa

È iscritto a parlare il senatore Molinari. Ne ha facoltà.

ma che non corrisponde alla realtà delle cose. Quindi, intervengo in modo assolutamente non polemico, perché anche nel confronto tra di noi che può e deve essere aspro, rimaniamo ai dati di fatto. ai dati di fatto. Se continuiamo a dire una cosa non vera non per questo diventa vera. Quando, cioè, si dice che questo Governo e la sua maggioranza hanno regalato 7,5 miliardi di euro alle banche, per chiunque ascolta ciò significa che lo Stato ha versato nelle casse delle banche 7,5 miliardi. Siccome questo non è vero, provo a dire che cos'è successo.

È solo una scrittura contabile interna, che sposta dalle riserve a capitale la somma indicata. Anche le banche detentrici delle quote effettuano una semplice scrittura contabile e rivalutano le loro quote, ma questa volta pagano le tasse sulla plusvalenza, senza aver intascato alcun soldo.

tali quote. Questo è quanto è avvenuto per adesso in alcuni casi e avverrà quando il processo sarà completato. Si può discutere

e comunque c'è un dato incontrovertibile: nel 2014 nessuno poteva onestamente, da un punto di vista intellettuale ed economico, dire che il capitale corretto per la Banca d'Italia fosse quello, come era allora, di 156.000 euro. Dico questo perché credo sia giusto, su questo terreno, un confronto sui dati. Ritorno adesso sul tema oggi in discussione, ripartendo intanto con il fornire alcuni dati fondamentali. Su cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo su una quota rilevante del sistema bancario italiano: le BCC e le Casse rurali sono 364, pari al 55,9 per cento del totale delle banche italiane. Stiamo parlando di 4.450 sportelli; di un patrimonio di 20,5 miliardi di euro; di 1.230.000 soci; di impieghi, nell'economia reale, per 135 miliardi e di una raccolta da clientela di 161,5 miliardi di euro. E questi sono dati al 30 giugno 2015.

Fondamentalmente, Barbagallo ha posto la seguente questione: esiste un problema di debolezza del modello di *governance* che produce, nell'attuale fase del mercato dei capitali, una difficoltà nel rafforzamento patrimoniale, che storicamente le BCC avevano risolto attraverso l'autofinanziamento, ma che l'erosione dei profitti dovuta alla crisi non consente più. il tema è il seguente: nel momento in cui, anche in considerazione delle nuove regole di vigilanza europea, il sistema delle BCC deve andare verso il mercato dei capitali, è necessario rafforzare il patrimonio ma, per far questo, occorre mettere mano all'intero sistema. C'è un altro dato fedele che ha spinto all'intervento, e cioè una maggiore vulnerabilità rispetto alla storia e alla tradizione molto lunga - in alcuni casi centenaria - delle BCC, quale deriva dall'aumento della quota dei cosiddetti crediti deteriorati, che in alcuni casi può essere derivata anche da *mala gestio*, o comunque da scelte bancarie sbagliate. Ma, più in generale, essa è frutto di un problema che le BCC hanno in considerazione, in realtà, di un pregio della loro attività, dato che più che altre banche - più di tante banche straniere, ad esempio - hanno un rapporto con l'economia reale. In sostanza, esse hanno dato soldi direttamente al sistema delle piccole e piccolissime imprese che hanno subito, in questa fase economica recessiva durata molto di più di tutte le altre crisi, un contraccolpo molto forte e quindi, conseguentemente, essendo più esposte, oggi hanno un aumento dei crediti deteriorati e hanno - dati Bankitalia - un tasso di copertura inferiore a quello del sistema. Quindi, rispetto alla domanda se si doveva o si poteva intervenire, al di là dello strumento, la risposta io credo che sia Ed è importante e apprezzabile - l'ho detto in Commissione e lo ripeto in Aula - il ruolo proattivo che Federcasse ha avuto in tutta questa fase con l'allestimento di un progetto di autoriforma. A differenza, per esempio, di Assopopolari e di quanto era accaduto per le banche popolari, Federcasse è riuscito a proporre al sistema, al Governo e alla Banca d'Italia un progetto di autoriforma.

cui, in estrema sintesi, le BCC non possono più continuare a svolgere attività bancaria se non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, la cosiddetta *holding*, che abbia un capitale di almeno un miliardo. Qui c'è un punto, però, su cui voglio essere chiaro: mentre era assolutamente condivisibile, ed è condivisa, l'impostazione data da Federcasse, e cioè l'idea del gruppo bancario cooperativo unico, della *holding*, del salto di qualità salto di qualità sia sul mercato dei capitali sia rispetto ai problemi - per esempio - di adeguamento e di *compliance* - è una risposta corretta - nel testo originario

Perché la *way out*? Io non sono ancora riuscito a trovare una risposta sul perché sia stata inserita la *way out* e sui termini con cui è stata inserita. Bisogna dare atto al Governo di avere ascoltato in parte, anche se non tutte, le critiche che sono state sollevate e nel lungo dibattito e nel confronto svolti in Commissione e in Aula alla Camera si è arrivati a un testo che presenta importanti revisioni: l'intangibilità delle riserve indivisibili, la possibilità di costituire i sottogruppi, la possibilità di scorporo dell'attività bancaria da parte della cooperativa con il pagamento della tassa del 20 per cento, confermando però la mutualità, e soprattutto con il parere obbligatorio di Bankitalia. Se ci fosse stata la possibilità di poter ancora ragionare e intervenire, credo che qualche ulteriore riflessione sul significato e sulle modalità della *way out* sarebbe stata auspicabile

delicati, siate intervenuti con la decretazione d'urgenza, mettendo insieme elementi eterogenei e una volta di più mortificando questo ramo del Parlamento, impedendoci, arriva con la fiducia incorporata, di apportare le necessarie correzioni (di alcune delle quali ha parlato il collega Fornaro), come nel caso delle cartolarizzazioni e della riforma delle BCC, in particolare. Su quest'ultima, nonostante l'importanza della posta in palio, siamo d'accordo anche noi che occorra e sia necessario intervenire, tant'è che i migliori auspici e le migliori aspettative avevamo trovato appunto nella alimentata autoriforma del credito cooperativo. nell'impianto che avete portato all'attenzione del Parlamento, tutto ciò sia stato tradito, perché avete partorito un pericoloso ibrido. Eppure, avevo apprezzato il progetto di autoriforma, per come ci era stato illustrato, tra l'altro, in un seminario tenuto al Senato. Ma quello che oggi ci volete propinare ha tradito quelle intenzioni, nate sotto i migliori auspici. Il primo obiettivo della riforma doveva essere salvaguardare la biodiversità del sistema creditizio, nel rispetto della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, anche nel nuovo mondo bancario che verrà a determinarsi dopo la BRRD e, quindi, l'introduzione del *bail in* (o proprio per quello). E invece ci si è dimenticati che l'obiettivo della banca cooperativa non è remunerare nel modo più elevato possibile il capitale, ma contribuire allo sviluppo economico della realtà locale, fatta

Che grave errore - come ha pure evidenziato il collega Fornaro - aver eliminato la possibilità di autorizzare fusioni e trasformazioni tra banche di credito cooperativo e banche popolari, lasciando come unica possibilità il solo ricorso alla forma di banca costituita in società per azioni. Il contratto di coesione tra le banche costituenti il gruppo doveva inoltre prevedere, indicando con esattezza i poteri attribuiti alla capogruppo (la cosiddetta *holding*), la disciplina della sua direzione e del suo coordinamento, ma nel rispetto delle finalità mutualistiche e della salvaguardia delle realtà locali, per l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e operativi necessari a tale attività. Il potere di controllo doveva solo avvenire in funzione dinamica ed essere mirato alla singola banca, per assicurarle il raggiungimento del consolidato contabile del gruppo, proprio a tutela degli interessi del territorio e degli utenti della banca medesima. Invece i poteri della capogruppo nei confronti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti, un'inusitata espansione del potere della capogruppo, che fa diventare ordinaria la facoltà della stessa di nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più dei loro componenti, facoltà originariamente prevista solo in casi eccezionali. Che l'esercizio di tale potere debba comunque essere motivato - così lo avete rappresentato - io credo che sia poca cosa, e a maggior ragione se quella motivazione non sarà puntuale, come avevo cercato di sostenere con un emendamento. L'intenzione, senz'altro apprezzabile, di voler rafforzare la competitività del gruppo e consolidarne la situazione patrimoniale sembra a maggior ragione venire meno quando poi viene estesa l'inapplicabilità delle disposizioni riguardanti la limitazione dell'acquisto di partecipazioni incrociate al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo, alle banche cui fanno capo cosiddetti sottogruppi territoriali, entità ibride che sono strutturalmente estranee alle classiche forme in cui si estrinseca lo scambio mutualistico di utilità. Possibile che non si intravede la pericolosità di una tale commistione? Non si prevede un compito facile - io credo - nella vigilanza che la Banca d'Italia dovrà operare sulla scorta delle disposizioni che la stessa sarà chiamata a dettare e sulla falsariga della regolamentazione che il Ministero dovrà emanare. E io spero che sia migliore di quella svolta in occasione delle ultimi crisi del settore, come quella di Banca Etruria *et similia*. In questo contesto di confusione tra i generi si innesta l'ampliamento del novero delle disposizioni che si potranno applicare alle banche di credito cooperativo, consentendo alle loro assemblee di nominare gli amministratori e alle società stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi, possibilità finora escluse dal codice civile; che, per le condizioni alle quali sono sottoposte, lasciano più di qualche dubbio sugli effetti concreti della loro gestione e utilizzo e sugli effetti combinati delle limitazioni della circolazione degli strumenti finanziari partecipativi e sulla modalità con cui vengono attribuiti ai loro possessori i voti in assemblea. Questo mette in crisi il principio del voto capitario, che è lo strumento con cui si è introdotto il metodo democratico all'interno di un settore più attento all'aspetto capitalistico che a quello sociale. Semmai il tentativo della riforma - io credo - doveva andare in direzione di scongiurarne la deriva personalistica e familistica del suo utilizzo - come avvenuto, ahimè, in alcune realtà locali - non eliminandolo però di fatto e favorendo, quindi, il capitale. Non dimentichiamo poi la possibilità che le azioni di finanziamento possono - così come le avete costruite - essere sottoscritte dalla capogruppo in deroga al vincolo di territorialità e ai limiti di partecipazione stabiliti per i soci ordinari, consentendone l'emissione - seppur sotto l'autorizzazione della Banca d'Italia - anche al di fuori dei casi di insufficienza patrimoniale e amministrazione straordinaria. Ma ciò che lascia davvero perplessi - e l'ha indicato anche il collega Fornaro -in questa tanto voluta quanto necessaria riforma è, così com'è stata costruita, la previsione del cosiddetto cosiddetto *way out*, che sancisce la possibilità di escludere l'effetto devolutivo, per come richiesto invece da una famosa pronuncia della Corte costituzionale nel 2008. Ora, in una formulazione che ha subito via, via modifiche, l'articolo 2 - nei commi che vanno dal 3-*bis* al 3*-quater* - esclude i predetti effetti devolutivi ove la banca di credito cooperativo coinvolta nelle predette operazioni straordinarie abbia un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, risultante dal bilancio al 31 dicembre 2015, sul quale il revisore contabile non abbia espresso rilievi - e meno male, vorrei dire - con l'unico onere - così lo avete costruito - di presentare alla Banca d'Italia un'istanza per conferire l'azienda a una società per azioni esercente attività bancaria All'atto del conferimento la banca verserà al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto come risultante dal bilancio. Quale sia - ripeto - il fondamento logico-giuridico di tale costruzione io non l'ho capito. Gli emendamenti che avevamo presentato, insieme agli altri amici, in Commissione per cercare di dare ordine in questo campo naturalmente sono stati rigettati, perché non possiamo toccare il pacco. tutto ciò avviene tacendo dell'altro grave problema operato in materia di cartolarizzazione dei crediti presente in questo provvedimento, ceduti dalle banche e dagli intermediari finanziari con sede in Italia e qualificati come crediti in sofferenza, per i quali si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia statale. La quantificazione forfettaria di tali coperture, infatti, rimane irrealisticamente pericolosa - mi permetta di dire, signor Vice Ministro - con l'ulteriore rischio che le disposizioni relative alla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, pur affrontando una problematica sistemica del settore, potrebbero implicare la diffusione di titoli tossici tra i risparmiatori che arriveranno da altre strade. Insomma, nello specifico sembra si sia persa un'altra occasione di smarcare il nostro sistema bancario da un modello unico; il nostro, contraddistinto da una struttura imprenditoriale formata essenzialmente da piccole e medie imprese, idonee per affrontare le sfide della flessibilità e dell'innovazione in campo internazionale, che avrebbe potuto e avrebbe dovuto trovare in questa riforma una nuova realtà di credito cooperativo. Il rischio è perdere la spinta di piccole ma importanti realtà che hanno contribuito, però, più delle grandi banche - e i dati ce li ha ricordati il collega Fornaro - a fornire credito alle piccole e medie imprese, ma anche ai consumi delle famiglie, sul territorio nazionale in questi duri anni di crisi. Il Paese gradirebbe sapere perché si sia voluto perdere quest'ulteriore occasione e, nel contempo, si sia voluto minare quel baluardo messo in Costituzione a difesa di concentrazioni nel settore finanziario e bancario, che deve invece mantenere una sua biodiversità. Non dovevamo rinunciare al disegno di una finanza partecipativa, in cui trovano posto sia i grandi che i piccoli e dove viene esaltato il principio democratico delle scelte. Il modello europeo di credito cooperativo che questa riforma mette seriamente a repentaglio è stato l'unico antidoto per contrastare lo strapotere dei grandi conglomerati finanziari e a maggior ragione oggi, in attesa di ritornare al modello di separazione che ha tenuto al riparo dagli effetti della crisi il sistema bancario, come quello canadese, che non lo ha mai abbandonato, in cui le banche commerciali (che accettano depositi e fanno prestiti) e le banche d'affari (che fanno emissione e negoziano titoli) sono separate. Speriamo - lo spero vivamente - che questa riforma non si tramuti nell'atto finale di un suicidio annunciato per il nostro settore bancario.

mi permetto di rivolgermi al Presidente del Senato, ai Capigruppo e a tutte le colleghe e i colleghi per porre un problema istituzionale. Vorrei sollevare un problema che mi sembra molto serio. Dal 2008 la vicenda Lehman Brothers ha scatenato e segnato l'inizio della crisi negli Stati Uniti d'America e in Europa. Le banche sono state protagoniste della crisi economica e ne sono state condizionate, perché naturalmente essa ha determinato in ciascuna un grande aumento delle sofferenze e, pertanto, ulteriori difficoltà nel poter elargire credito.

di approvare la delega e di non far andare perso il lavoro realizzato nella precedente legislatura sia alla Camera che al Senato.

il Senato della Repubblica italiano non ha concretamente potuto occuparsi dei problemi del sistema bancario italiano. Questa è la verità.

Poi c'è stata la vicenda delle quattro banche, che è stata affrontata in un emendamento presentato alla Camera alla legge di stabilità

abbiamo con fatica letto il provvedimento. Adesso arriva il provvedimento delle BCC. Con correttezza e lealtà, delle quali voglio dargli atto, il vice ministro Morando in 6a Commissione ha ha detto con molta chiarezza che il Governo cercava di operare affinché il testo della Camera non fosse modificato dal Senato. E questa è stata la filosofia con cui il provvedimento è stato approvato. La Camera lo aveva esaminato, ma noi non abbiamo la possibilità di esprimerci concretamente. Per la verità, in Commissione abbiamo almeno approvato quattro o cinque ordini del giorno. Questo è il contributo che abbiamo dato. sarà sottoposta a *referendum* se la Camera, com'è prevedibile, l'approverà e gli italiani si pronunceranno, e poi sarà applicata dalla prossima legislatura. Mi rivolgo con molta energia e prego il vice presidente Gasparri di trasmettere il senso di questo intervento al presidente Grasso. Mi rivolgo al presidente Grasso, agli stessi Presidenti dei Gruppi, a tutti senatori perché una situazione di questo genere è inaccettabile sul piano istituzionale. Per quanto riguarda il merito del provvedimento,

alle numerose osservazioni che le Commissioni 10a e 14a, nel dare parere non ostativo, hanno formulato in proposito.

fatto. Concludo rivolgendo per l'ennesima volta al presidente Grasso un appello: per favore, tuteli il ruolo del Senato.

Signor Presidente, all'attenzione di quest'Assemblea è arrivato un altro pezzo importante dell'intervento che il Governo intende esperire sul sistema bancario, iniziato iniziato l'anno scorso con la riforma delle banche popolari, una misura che nelle intenzioni avrebbe dovuto razionalizzare un comparto, ma che nei fatti si sta rivelando il salvataggio di qualcuno in difficoltà. Lo stesso spirito ha accompagnato l'adozione, a fine 2015, di un'altra normativa talmente urgente e necessaria da essere traslata nella legge di stabilità. Mi riferisco al cosiddetto salva banche, balzato agli onori delle cronache più per le questioni familistiche legate a una delle quattro banche interessate dal provvedimento che per l'operatività di quella stessa banca.

Il salva banche è un provvedimento claudicante, in bilico tra le novità del *bail in* e i tradizionali aiuti di Stato, che ha portato a un braccio di ferro con la Commissione europea. L'Unione europea ancora non ha dato il proprio via libera alle modalità con le quali l'Esecutivo intende risarcire le vittime di quella operatività e che ha reso necessario il decreto-legge che stiamo ora esaminando, contenente interventi necessari a fronteggiare gli effetti nefasti della crisi. Primo fra tutti è lo sviluppo del mercato dei cosiddetti *non performing loans* (NPL), uno *stock* gigantesco di crediti deteriorati, accumulato negli anni, che costituisce il vero freno da la scarsa offerta di credito all'economia da parte delle banche. Per i crediti deteriorati è previsto l'intervento dello Stato, attraverso un'apposita garanzia che, tuttavia, non appare adeguata all'obiettivo prefissato. Sebbene sia il frutto anch'essa di una "negoziazione" con la Commissione europea, salutata positivamente dal Governo, questa garanzia a noi Conservatori e Riformisti sembra caratterizzata da elementi che destano diverse perplessità. se raggiungerà il suo scopo una garanzia, che tra l'altro è prevista solo sui titoli cosiddetti *senior* (ovvero più sicuri), che diviene efficace solo dopo che la banca abbia trasferito il 50 per cento più 1 dei titoli cosiddetti *iunior* (ovvero quelli più rischiosi). Mi chiedo inoltre se le risorse pubbliche destinate a questo intervento siano state previste adeguatamente, o se corriamo il rischio, per noi molto concreto, di trovarci a breve - magari il prossimo anno - a dover intervenire per rimpinguare la somma oggi messa a disposizione, data la possibilità di estendere quella garanzia. Quello all'esame dell'Assemblea è certamente un provvedimento composito e complesso, che costituisce altresì il veicolo per la riforma di un pezzo importante del settore creditizio: il credito cooperativo. Qui è una buona parte della storia economica del Paese a essere investita dalla proposta del Governo. Quella alla nostra attenzione è, infatti, la terza fase della storia del credito mutualistico in Italia. Lo ricordiamo soltanto per rendere omaggio a quei pionieri che, circa un secolo fa, inventarono formule locali e più antropologicamente confacenti alla cultura e alle esigenze contadine insite nella società dell'epoca, espressione delle piccole e medie comunità regionali e provinciali. Il lavoro, la fatica, la propensione e l'educazione al risparmio, l'uso mutualistico del denaro, in quel periodo storico, sono alla base del fenomeno virtuoso delle casse rurali e artigiane. Le casse rurali rappresentano la prima fase; la seconda è costituita dalle trasformazione intervenuta nel 1993 in banche di credito cooperativo. Ora siamo alla terza fase, quella della *holding*, ovvero la formazione del terzo gruppo bancario italiano, che è auspicabile possa avere effetti positivi sull'economia dei territori. infatti, assolutamente importante che il credito cooperativo continui a servire gli operatori economici, gli imprenditori piccoli e medi e le famiglie della multiforme provincia italiana. Ci congratuliamo con il sistema istituzionale delle BCC, perché ha saputo conservare le sue prerogative e ha difeso a denti stretti le peculiarità di fare credito e di normarlo, a cominciare dal basso. Questa, infine, è una riforma che parte dal basso e, cioè, dai diretti portatori di interessi. È una riforma complessa, partita con il piede sbagliato: penso solo al testo originario, in cui mancava la possibilità di recedere dalla *holding* e che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata in qualche modo aggiustata. interventi che hanno delineato una nuova operatività, che può essere valutata positivamente per un solo motivo: la salvaguardia della diversità, che comporta la compresenza sul mercato di una parte importante della storia e della cultura solidaristica e mutualista del credito del nostro Paese. In conclusione, il capitalismo di oggi appare camaleontico e onnivoro, recepisce e assorbe valori, simboli e parole della società civile e della politica. Il credito cooperativo resta un baluardo di tutto ciò. Mutuando un titolo contenuto nell'*house organ* di Federcasse, la Federazione delle banche di credito cooperativo, ricordo che «l'economia che è solo economia diventa diseconomia». Diventa, in buona sostanza, tritacarne, umiliazione, cinismo. Mortifica gli uomini e le donne che intraprendono, che rischiano, che mettono a capitale il proprio lavoro, evocando la crisi dei valori e dei fondamentali della società italiana. Pertanto, auspichiamo che questa riforma contribuisca a creare valori. PRESIDENTE. È

particolare con il *bail in -* anche sulle raccolte per gli stessi istituti di credito. Lo strumento legislativo previsto in Costituzione per le situazioni di straordinaria necessità e urgenza viene impropriamente utilizzato in una riforma dell'intero sistema del credito cooperativo, che rappresenta una quota consistente del sistema creditizio italiano; un sistema complesso e articolato, avente più di centotrenta anni di storia, formato da 364 banche radicate capillarmente nel territorio, con oltre 1,2 milioni di soci, 37.000 dipendenti e oltre 6 milioni di utenti; un grande patrimonio che promuove la solidarietà, sociale e intergenerazionale, attraverso istituti di credito ispirati ai principi dell'assistenza mutualistica. Come si può parlare di urgenza di una riforma per una realtà così diffusa? Certo, ci sono criticità che presentano rischi di insolvenza, ma riguardano meno di 20 BCC sul totale, che si potevano trattare a parte. Anziché procedere con un normale *iter* legislativo che risalta il ruolo al Parlamento, il Governo non solo ha scelto uno strumento sbagliato, che comprime tempi e dialoghi e imbavaglia il Senato nell'ennesima fiducia. Nello scrivere il provvedimento ha anche dimostrato la sua inadeguatezza. pieno di innesti e rimandi a norme esistenti, con contraddizioni, opacità, indeterminazioni che creano confusione e dubbi interpretativi per chi queste leggi le deve applicare. Non solo: anche qui si ritrova il marchio di fabbrica renziano, che è la cura non dell'interesse collettivo, ma di una ristretta cerchia di parenti, amici e sodali, che condizionano e stravolgono le leggi a proprio beneficio. Dopo Banca Etruria e Tempa Rossa, anche in questo decreto-legge non è mancato l'intervento di un membro del Governo, riconducibile al giglio magico, che ha forzato la mano con l'introduzione della l'introduzione della famosa clausola del *way out*. II Governo Renzi, in fase di conversione del decreto-legge alla Camera, si è inventato una scappatoia per gli amici che non gradivano l'obbligo di aderire al gruppo bancario unico; una norma che, in spregio all'articolo 3 della Costituzione, è stata tagliata su misura per le banche toscane amiche, come la BCC di Cambiano, guidata da papà Lotti, oppure ChiantiBanca, la ex banca di Denis Verdini, oggi soccorritore della maggioranza. Quella che si è palesata è un'imbarazzante difesa del territorio toscano, con cifre studiate a tavolino! Parlo di imbarazzo, perché tale si è manifestato tra gli esponenti di maggioranza e Governo, che in Commissione non avevano un argomento plausibile nella difesa della clausola scappatoia. Scusate ma, se il Governo ha posto l'asticella a un miliardo per il gruppo bancario cooperativo, come può la soglia patrimoniale di 200 milioni, la cosiddetta scappatoia, considerarsi di tutta sicurezza per una banca che opera nella forma di SpA? Sottolineiamo come questo provvedimento conferma l'incapacità della maggioranza e della sinistra di valorizzare modelli socioeconomici che ci sono propri e naturali e, dunque, la volontà di inseguire quelli che non ci appartengono. L'Italia è un insieme di territori, culture, lingue e comunità diverse. E in questa varietà e specificità del nostro Paese, è vero che a volte trovano spazio eccessi e limiti del localismo, ma sono radicate anche le nostre immense risorse. Con questa riforma siamo lontani dal superare questi limiti. Il nuovo gruppo bancario cooperativo non si avvicinerà minimamente, in dimensione, a gruppi omologhi presenti in Francia, Germania o anche nella piccola Olanda. Improbabile dunque che si ottenga il risultato di creare una *holding* italiana del credito cooperativo che possa confrontarsi ad armi pari con analoghe presenti sul mercato internazionale. In compenso, si rischia concretamente di perdere definitivamente un patrimonio fatto di aziende di credito cooperativo fortemente radicate nel territorio, in simbiosi stretta con le diverse realtà economiche e produttive del Paese. Peccato che il decreto-legge riconosce queste specificità alle sole Province autonome di Bolzano e Trento, ma le ignora nel resto del Paese, quando sono invece di tutta evidenza. hanno sempre adattato, nella stragrande maggioranza dei casi con pieno successo, il loro modello di finanziamento alle diverse realtà in cui operavano: un sistema peculiare che ha dimostrato una straordinaria capacità di resistere e ammortizzare gli effetti di crisi finanziarie devastanti come quella vissuta nel 2008, con code anche negli anni seguenti, e in molti casi le banche di credito cooperativo - lo ricordo e sottolineo - sono rimasti gli unici istituti ad erogare il credito a famiglie e imprese. Con la precipitosa riforma che votiamo oggi rischiamo seriamente di perdere un patrimonio di valore inestimabile per l'incapacità dimostrata da questo Governo di riconoscerlo, valorizzarlo ed apprezzarlo. Noi riteniamo che il decreto-legge, per fare spazio alle ragioni del libero mercato, reca con sé degli aspetti pericolosi, per cui il carattere di mutualità, la cooperazione e altri valori rischiano di essere distrutti. Sia chiara una cosa: se pensate di rilanciare l'economia del Paese, in seria difficoltà, continuando a propinare modelli che privilegino le grandi realtà, tra grosse banche, grosse società stile FIAT, grandi Comuni, frutto di fusioni imposte dall'alto, siete fuori strada. Fermatevi prima di andare a sbattere e di far sbattere il Paese. Non dimenticate - lo ribadisco - che questo Paese ha una storia di successo che si è retta soprattutto grazie ad un sistema economico, produttivo e sociale basato sulla piccola e media impresa, sugli instancabili artigiani, sui commercianti, e grazie ad un sistema di credito capillare che ha funzionato come supporto e rete di sicurezza. I tempi cambiano, ma di loro c'è sempre bisogno. ogni modo, la partita vera di questa riforma, che determinerà la reale portata e gli effetti della stessa, si giocherà con il lavoro che sarà fatto nei prossimi due anni. Se i patti e il contratto di coesione non saranno scritti direttamente dalle ma esclusivamente da Bankitalia o dal gruppo bancario cooperativo, ci saranno gravi ripercussioni sul territorio. Faccio solo un esempio. Se emergerà la volontà di fare una centrale unica di acquisto avremo la conferma che i nostri dubbi sono fondati in ordine alla sottointesa volontà di distruggere le economie locali. Mi avvio alle conclusioni ricordando a Renzi e ai membri del Governo, a proposito di banche, che ci sono ancora decine di migliaia di persone che attendono da tempo risposte. Sono quei risparmiatori che prima sono stati ingannati da Banca Etruria, Banca delle Marche, Carichieti e Cariferrara a sottoscrivere obbligazioni subordinate spazzatura, e che poi dallo scorso novembre sono stati truffati dal Governo con il decreto salva banche, che ha fatto perdere loro i risparmi di una vita. Un provvedimento pessimo, poi confluito nella legge di stabilità che solo a seguito di proteste che hanno visto in prima fila la Lega Nord a fianco dei risparmiatori ha istituito un fondo di ristoro di 100 milioni, ancorché decisamente insufficiente, ma che al contempo ha introdotto l'arbitrato e relativi criteri, cioè elementi discrezionali pericolosi che scontenteranno tutti e daranno certamente luogo a contenziosi. Avevate promesso ai risparmiatori una corsia accelerata per chiudere la partita dei ristori entro la fine di gennaio; promessa disattesa. Poi avete ipotizzato un aumento del fondo a 280-300 milioni, per restituire integralmente il furto esercitato con destrezza; solo chiacchiere. Intanto, il 30 marzo, termine fissato per legge per l'emanazione sia del decreto ministeriale che doveva stabilire i criteri per l'arbitrato, sia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la scelta degli arbitri, è stato abbondantemente superato. È assurdo: bastonate gli italiani se violano le leggi, se ritardano di pagare una delle sterminate tasse e poi voi fate peggio. Vergogna! Anche in questa occasione state dimostrando di essere un Esecutivo fallimentare e inaffidabile, che dunque deve andare assolutamente a casa, perché non solo non sa risolvere i problemi degli italiani, ma addirittura in molti casi li aggrava. Sto parlando della subalternità del nostro Paese all'Europa, alla Turchia, all'India, all'Egitto; delle tasse che non calano e degli studi di settore vessatori. Sto parlando del lavoro e della disoccupazione, che dopo la deroga della decontribuzione sulle assunzioni sta ancora aumentando. Sto parlando del debito pubblico accresciuto per manovre finanziarie dal sapore elettorale, dell'insicurezza dei territori e della gestione scellerata dell'immigrazione clandestina; una bomba che quest'anno deflagrerà. No, signor Presidente, non ci siamo assolutamente; il bene comune avrebbe voluto tutt'altra cosa che non questo decreto-legge. MPL))*. Signor Presidente, gentili colleghi, il provvedimento di cui stiamo discutendo oggi all'interno di quest'Aula sarebbe un esempio lampante da seguire in materia di regolazione bancaria. Si tratta di un grande esempio di riforma dal momento che alla redazione del testo ha partecipato attivamente Federcasse e, dunque, molti istituti del credito cooperativo. Sarebbe auspicabile utilizzare queste modalità di redazione dei testi in molte più occasioni e su molte delle materie su cui quest'Assemblea è chiamata ad assolvere la sua funzione principe, quella legislativa, della quale, però, con riferimento al provvedimento in oggetto, mi sembra si sia palesemente abusato. Dico questo dopo un'attenta lettura dell'articolato, il quale fornisce una disciplina così dettagliata da risultare patologica. Cari colleghi, consentitemi di dire che probabilmente ci troviamo di fronte ad uno degli interventi più dirigisti che sia mai stato fatto in campo economico e nel campo della regolazione bancaria. Ci si è lamentati periodicamente delle regole che l'Unione europea, attraverso direttive e regolamenti, ha imposto negli ultimi anni al sistema bancario italiano, vincolandolo rigidamente a specifici parametri, e noi oggi ci troviamo a discutere un provvedimento che riesce nella pessima impresa di superare il dirigismo europeo in materia economica e bancaria. L'idea, alla base della riforma, che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo sia consentito solo agli istituti cooperativi che siano parte di un più grande gruppo bancario cooperativo, al quale hanno deciso di aggregarsi, ha come potenziale conseguenza la fine del credito cooperativo in Italia, mentre in altri Paesi, come la Germania, il Belgio e la Svezia, le forze politiche, economiche e sindacali lottano senza tregua per difendere le proprie banche cooperative. Infatti, l'aggregazione delle BCC in grandi gruppi bancari cooperativi non fa altro che snaturare l'aspetto locale delle stesse BCC, che della territorialità hanno fatto un tratto distintivo nonché un loro punto di forza. Ciò danneggerà le aree più deboli del Paese, soprattutto il Mezzogiorno, dove le banche del credito cooperativo rappresentano da sempre un esempio d'intermediazione finanziaria del e sul territorio, proprio in virtù della loro autonomia che gli ha consentito, storicamente, di essere più vicine e più attente alle esigenze dei clienti, che si trattasse di semplici cittadini o di imprese. Quelle stesse imprese che oggi, per il combinato disposto della recessione e del livello di regolazione, difficilmente riescono a trovare interlocutori finanziari disposti a dare loro fiducia. All'interno di quest'Assemblea rappresento con orgoglio quella Regione italiana che, stando alle ultime rilevazioni ISTAT, è l'ultima per reddito medio dichiarato. Ovviamente mi riferisco alla Calabria, la stretta sul credito, dovuta alla congiuntura economica ed al radicato pregiudizio dei principali istituti di credito italiani, ha avuto pesanti ripercussioni per tutto quel mondo imprenditoriale che di essa dovrebbe essere il primo motore, e che è tristemente destinato all'oblio. Una maggiore attenzione alle dinamiche locali da parte del Governo avrebbe probabilmente favorito l'adozione di un provvedimento che non snaturasse, in modo così prepotente, la natura stessa del credito cooperativo. Si sarebbe potuto imboccare il percorso di una razionalizzazione delle BCC su base regionale, invece si è voluto percorrere ostinatamente il sentiero di una riforma che cancellerà la tipologia cooperativa nel sistema bancario, riducendo i margini di concorrenza e di competitività. Non si può dimenticare che il nostro Paese ha fondato la sua storia economica e finanziaria su una differenza fondamentale: quella fra grandi banche e piccole banche. Con il decreto-legge che questo Parlamento si accinge a convertire, questa distinzione si appresta nei fatti a scomparire. E non è tutto: il cosiddetto fardello regolatorio si estende dalle grandi banche alle piccole, con un aumento inevitabile delle regole che i piccoli istituti di credito cooperativo saranno chiamati a rispettare. Aumenteranno le rigidità, le regole e le limitazioni al credito che da tempo le imprese e le famiglie delle aree più deboli del Paese stanno sperimentando. Assisteremo alla fine delle banche del territorio, un tempo vero e proprio fattore di sviluppo,

In nome dell'efficienza bancaria, perderemo in accumulazione di capitale sociale, di cui il credito cooperativo è straordinario generatore. Avremmo appoggiato con convinzione veri obiettivi di razionalizzazione dei sistema del credito cooperativo, quale la riduzione del 50 per cento del numero delle BCC nel giro di cinque anni (da 400 a 200). Avremmo gradito una partecipazione dei gruppi bancari più grandi nel capitale delle BCC, al fine di rafforzarle e renderle competitive sul mercato bancario, ma sempre mantenendo la maggioranza del capitale nelle mani delle Si è preferito invece optare per uno spiccato interventismo dello Stato nel sistema bancario, interventismo che non fa altro che sfumare, fino a farle divenire impercettibili, le buone intenzioni di efficientamento del sistema del credito cooperativo alla base del provvedimento, del quale, cari colleghi, credo di avervi espresso alcune preoccupanti criticità. Signor Presidente, senatrici e senatori, signor Vice Ministro, l'Assemblea del Senato si ritrova ad affrontare un tema che è stato ed è oggetto di grande attenzione da parte dell'opinione pubblica. La vicenda delle quattro banche fallite, la necessità di offrire maggiori tutele ai risparmiatori, le nuove regole europee sul *bail in* e le oscillazioni in borsa che hanno riguardato il Monte dei Paschi di Siena e altri istituti bancari impongono al nostro sistema di dotarsi

di un territorio in passato tra i più poveri d'Italia e che, ancora oggi, costituisce un fondamentale punto di riferimento per il tessuto imprenditoriale, per le famiglie e per il volontariato. Perché il credito cooperativo, con il suo radicamento, ha favorito la coesione sociale e svolge ancora oggi una funzione di supplenza su tutta una serie di servizi in quelle località in cui sono venuti meno uffici postali ed altri servizi essenziali. Per dare la giusta dimensione, basta guardare i numeri: in Trentino, su una popolazione di 537.000 abitanti, il credito cooperativo vanta 127.000 soci, quasi 3.000 dipendenti, 41 casse rurali e 365 sportelli distribuiti in tutto il territorio provinciale. Il 28 per cento della popolazione sopra i diciotto anni è socio, cento delle famiglie trentine ha fatto ricorso ad un credito erogato dalle casse rurali, così come il 50 per cento delle aziende. le casse rurali trentine coprono quasi il 50 per cento dei finanziamenti alle imprese e il 64 per cento di quelli alle famiglie. Il distretto del credito cooperativo trentino, negli ultimi sei anni, ha versato allo Stato 1.066 milioni di euro di imposte ed ha devoluto, tra il 2009 e il 2014, più di 115 milioni di euro per interventi sociali a favore della comunità, che hanno interessato la cultura, la scuola e la formazione, i giovani, lo sport e l'assistenza. Inoltre, la tutela dei risparmiatori è una questione che in Trentino è stata posta ben quarantadue anni fa, con la nascita, nel febbraio del 1974, della Cassa centrale delle casse rurali trentine SpA, che raccoglieva le 133 casse rurali allora operanti, proprio per far fronte alle difficoltà che le singole casse avrebbero potuto incontrare. Da allora, tutte le crisi del credito trentino sono state coperte e ammortizzate dalla Cassa centrale, che non ha mai pesato sulle altre realtà del credito cooperativo italiano. Questa lunga premessa, colleghi, mi è parsa doverosa non tanto per esaltare il sistema del Trentino-Alto Adige/Südtirol quanto per evidenziare a quest'Aula, e al Governo in particolare, che laddove c'è una realtà con tradizioni consolidate di buon funzionamento del sistema, bisogna intervenire con grande cautela. Le casse rurali del Trentino e la Cassa centrale, come ho ribadito a novembre in una lunga lettera al ministro Padoan, hanno pagato un prezzo altissimo per il salvataggio delle quattro banche: ben 25 milioni di euro versati nel giro di pochi giorni. Pur capendo le ragioni del Governo, non nascondo che quel provvedimento è stato per noi motivo di grande sofferenza per il modo in cui è intervenuto su un sistema come quello trentino che ha una sua forte specificità e che da sempre costituisce uno dei capisaldi della nostra autonomia. Qui non vogliamo mettere in discussione il principio sacrosanto per cui andavano tutelati i correntisti delle quattro banche, quanto la modalità con cui tutto questo si è concretizzato. sottolineo il fatto che le casse rurali trentine non potranno ricorrere, un domani, al fondo nazionale, non essendo riconosciute, per la ridotta dimensione, come banche di interesse pubblico. anche l'entità degli importi richiesti. Vi sono istituti che registravano perdite di 10 milioni di euro cui è stato chiesto un milione per il salvataggio delle altre quattro. E ve ne sono altri che erano in attivo e che sono finiti in perdita con la situazione, davvero paradossale, che adesso tutte sono chiamate a un nuovo intervento a livello locale per aiutare quelle casse rurali che, con l'esborso di fine anno, sono andate in difficoltà. Mi auguro davvero che una situazione così ingiusta non si ripeta più. Allo stesso tempo, ci sembra doveroso sottolineare che, nel suo impianto complessivo, il decreto-legge in conversione, per come è stato corretto, ha comunque il merito di tenere conto della specificità del sistema italiano, evitando contaminazioni con modelli come quello francese e olandese, che poco hanno a che fare con le necessità del nostro credito. che è stata introdotta una norma a tutela dell'indivisibilità del patrimonio di quelle banche di credito cooperativo che intendono affidare la loro attività bancaria a una società per azioni. Così come riteniamo che siano state fissate soglie abbastanza ragionevoli per la costituzione del gruppo o dei gruppi bancari cooperativi in merito all'uscita dal sistema per quelle banche che, avendo 200 milioni di patrimonio, intendono intraprendere questa strada. Sottolineo anche la norma dei sottogruppi territoriali che rispecchiano e valorizzano le presenze cooperative rilevanti che operano sul territorio nazionale, consentendo di organizzare vasti ambiti di territorio senza ledere l'impianto organico facente capo alla *holding*, in quanto i sottogruppi territoriali sono tenuti a partecipare ad essa. Tuttavia, a proposito della capogruppo, la confluenza di 365 istituti di credito - che hanno per loro natura scopo mutualistico - in una *holding* con natura giuridica di società per azioni, suscita qualche perplessità. Per questo ci pare di estrema importanza il fatto che siano inserite nello statuto della capogruppo apposite clausole di garanzia per la tutela dello scopo mutualistico che sta in capo alle banche di credito cooperativo che ad essa aderiscono. L'opportunità di attrarre capitali esteri sia dentro che fuori il movimento cooperativo in una *holding*-capogruppo, che per il 51 per cento resta comunque in mano alle banche di credito cooperativo, va considerato un processo evolutivo per consentire e favorire l'accesso al mercato dei capitali di rischio ed il rafforzamento patrimoniale. In questo contesto possono anche delinearsi profili di rischio per i risparmiatori, quando l'apertura al mercato viene fatta senza rispetto del principio di sana e prudente gestione. La cosiddetta *way out* riteniamo sia un istituto non degno del sistema cooperativo. È francamente un errore che si poteva evitare, come hanno detto anche altri colleghi poco fa. Le correzioni che ci sono state mitigano, ma non risolvono del tutto il problema. Un altro aspetto che ci sta particolarmente a cuore e sul quale sarà importante intervenire è il poter prevedere che i benefici fiscali dell'attività svolta dalle casse rurali rimangano sul territorio di cui sono diretta espressione. Non è possibile immaginare una configurazione diversa in quanto verrebbero depauperate proprio quelle comunità e quei territori che producono ricchezza, con lo sforzo di tutti i clienti e di tutti i soci. Come ho già detto, prendiamo atto delle significative correzioni che sono state apportate, e qui devo rendere merito al vice ministro Morando che se ne è fatto carico. Ma rimaniamo assolutamente convinti, e i dati storici di bilancio sono lì a confermare la validità della nostra posizione, che era molto meglio, al dì là della configurazione dei territori su cui operano, consentire ai gruppi che hanno mostrato stabilità economica di poter mantenere la loro autonomia operativa, anziché metterli sotto un unico cappello nazionale. Come autonomisti, come istituzioni locali e come delegazione parlamentare ci siamo mossi in maniera compatta e in sintonia con il credito cooperativo, riuscendo a ottenere significativi risultati, come quello che, all'articolo 37-*bis* di modifica del testo unico bancario, prevede per le banche di credito cooperativo delle Province autonome la possibilità di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi, così come la possibilità che il Ministro possa stabilire le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Quello che vorrei far capire a quest'Aula è che nel nostro territorio il sistema cooperativo - come ho avuto modo di sperimentare personalmente anche durante il mio mandato di assessore provinciale e regionale alla cooperazione e al credito costituisce una delle caratteristiche peculiari del nostro essere autonomi. Che si tratti del mondo agricolo, del sistema sociale, del consumo o del credito, il poter disporre di un sistema che coinvolge direttamente le persone, le famiglie e le imprese e le responsabilizza in tutti i campi della vita economica e sociale non può essere considerato né un'anomalia, né un fastidio da eliminare, ma deve essere visto invece come una grande risorsa e come un modello da assumere per il resto d'Italia. Per questo, ogni volta che vengono intaccati i principi che sono alla base di questo sistema, noi siamo preoccupati e rivendichiamo la bontà della nostra storia e la validità del nostro modello. Il mio auspicio è quindi che gli impegni politici assunti dall'Esecutivo, anche attraverso l'accoglimento di alcuni emendamenti e delle sollecitazioni della delegazione parlamentare del Trentino-Alto Adige/Südtirol, siano rispettati e che ai sottogruppi territoriali possa essere riconosciuto il giusto grado di autonomia. Ringrazio in particolare il vice ministro Morando, ma anche il sottosegretario Baretta, che hanno ascoltato le nostre sollecitazioni e che - in particolare il Vice Ministro - in parte le hanno recepite. Credo che l'obiettivo debba essere quello di un sistema solido, sufficientemente patrimonializzato, che intenda la tutela del risparmio come mantenimento di un forte legame con il territorio e - consentitemi - anche una forte dimostrazione di democrazia, perché le casse rurali e le banche di credito cooperativo sono comunque gestite dai soci e ogni testa vale un voto. Il credito cooperativo è nato anche per svolgere una funzione di carattere sociale e a questa sua missione deve essere sempre ricondotto, pena la perdita di un patrimonio di valori, di responsabilità e di protagonismo dei territori, ai quali sarebbe assurdo dover rinunciare.

Da questo dobbiamo partire, perché, se dovessimo fare un intervento in discussione generale in ragione della discussione degli emendamenti e quindi anche del possibile accoglimento dei migliorativi da noi proposti, tenteremmo di spiegare quali sono i contenuti degli emendamenti, perché chiediamo quelle modifiche e che finalità esse hanno. Invece, siccome questa possibilità non c'è, o facciamo, come alcuni, un intervento di ringraziamento, oppure facciamo, come altri, un intervento di critica. Questo lo dico perché ho una qualche difficoltà. Non penso che questo provvedimento sia pessimo: penso che abbia aspetti certamente utili, che sono stati anche richiesti dai soggetti interessati e dal sistema della cooperazione; che costruire una dimensione più ampia sia funzionale ad aumentare capacità di stare sul mercato, soprattutto a sostegno della impresa e della piccola e media impresa presente sul territorio, in settori sicuramente importanti come quello dell'artigianato, dell'organizzazione dei servizi e dell'agricoltura; versi, abbia grandi limiti sul piano della solidità del sistema individuato, soprattutto in ragione del cosiddetto *way out*, ovverosia della possibilità di uscita (credo che questa sia una critica che stava a fondamento di alcuni tentativi di correzione che si volevano portare anche in Senato). Ciò detto, rimane una questione che è davanti agli occhi di tutti noi: la scelta di operare per capitoli, non avendo il quadro del testo. Noi affrontiamo il tema del risparmio e del credito - perché il sistema finanziario ha questi due capisaldi capisaldi - con capitoli a se stanti, come se dovessimo costruire un sistema con parti stagne. il sistema finanziario del risparmio e del credito è unico, ha una sua unicità; si articola in modo differente, agisce sul mercato in modo differente, ha riferimenti culturali e sociali anche diversi, ma è un uno, un unico sistema. Siccome è così, noi ci saremmo aspettati che i provvedimenti che sono oggi all'attenzione, di volta in volta promossi con decreti-legge con carattere di urgenza, fossero invece stati oggetto di un'iniziativa, magari del Governo, organica. Badate: la distanza, anche temporale, tra un provvedimento e l'altro non è così grande da non rendere da non rendere possibile la strada più trasparente e più coerente di un provvedimento unico, articolato per ogni aspetto in modo efficace e tale da consentire anche una comprensione più diretta, non solo da parte degli addetti ai lavori, ma soprattutto da parte dei cittadini. I cittadini

Il risparmio, il deposito e le disponibilità delle banche e del sistema finanziario sono fatti dai contributi sistematici dei cittadini, dei cittadini lavoratori

perché alimenta sospetti, crea dubbi, avanza la possibilità che siano formulate perplessità da parte di soggetti, anche non nazionali, anche stranieri, che hanno interesse a indebolire il nostro sistema finanziario. È di questi giorni chiamare - fitta e sistematica critica che viene sulla solidità del sistema bancario nazionale

internazionali. Proprio per questa ragione e per tutte le vicende che hanno preceduto questo e altri provvedimenti che si sono dovuti adottare (o che hanno seguito altri provvedimenti che si sono adottati), avere il coraggio di dire: questa è la norma quadro, questa è la cornice dentro cui ci muoviamo, magari anche

di ciò i cittadini e neppure i soggetti che più sono vicini a quegli istituti di credito,

il nostro sistema finanziario deve assumere questa dimensione e avere queste qualità; questi sono i soggetti che stanno in campo; per questo tipo tipo di soggetti sono previste queste particolari possibilità, per altri queste altre; le regole di controllo, verifica

perché le banche sono le depositarie di tutti i nostri risparmi e anche di tutti i nostri depositi

magari con un altro provvedimento che - spero - questa volta non abbia la forma della decretazione d'urgenza e con la possibilità di un voto che - spero - non sarà di fiducia,

Tante volte in questa Aula ci siamo ritrovati a parlare di ambiente e sicurezza del territorio. Sono temi che so che questo Governo ha nella sua agenda e che, anche grazie al contributo del ministro Galletti, ritiene di fondamentale importanza. Da quest'Assemblea oggi voglio lanciare un SOS che riguarda l'ecosistema fluviale del Brenta, in Veneto, in un territorio compreso in diversi Comuni del Padovano, tra cui Carmignano di Brenta, Fontaniva, Cittadella e molti altri.

Nei cantieri si sta procedendo a una riduzione di superficie forestale in aree con vincolo idraulico. Stanno tagliando le piante per poi procedere, in una seconda fase, con i lavori per la realizzazione dei pozzi. Ho chiesto al Ministro dell'ambiente - cui ho presentato in queste ore un'interrogazione parlamentare - che il Governo prenda una posizione chiara sulla vicenda, considerando che questi lavori sono partiti ignorando un accordo di programma e, soprattutto, considerando che con un decreto la Regione ha escluso in autonomia qualsiasi eventuale verifica in termini di valutazione di impatto ambientale, essendo il fiume Brenta di competenza nazionale. Le preoccupazioni espresse da cittadini e amministratori locali e le critiche

alla Regione di non macchiarsi di un intervento così invasivo, che rischia seriamente di devastare, dal punto di vista ambientale, il fiume Brenta. Ho chiesto al ministro Galletti e al Governo innanzitutto se siano a conoscenza di tali problematiche e se non ritengano opportuno intervenire nelle sedi competenti, mettendo in atto azioni utili alla salvaguardia di un ecosistema così importante. Difendiamo il Brenta, difendiamo il nostro fiume! Il Governo fermi una vera e propria opera di devastazione ambientale.